Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

il caso del momento segnato dalla discussione del disegno di legge recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Lo devo ringraziare anche per aver sopportato in maniera oserei dire stoica gli attacchi, che io definisco vergognosi, da parte di tutto quell'apparato mediatico che si è venuto a costruire attorno alla discussione di questo

Probabilmente questi contenuti non sono stati nemmeno affrontati da parte di chi guadagna con i *follower* e con i *post* su Facebook e Instagram, ma non voglio neanche degnare di troppa attenzione queste persone perché a noi interessa il merito di questo provvedimento, a differenza - ripeto - di quanto è stato detto anche in questa Aula nella giornata di ieri e nelle giornate

abbiamo voluto portare al centro il contenuto, ma per affrontare il contenuto di un provvedimento di questo tipo abbiamo correttamente richiesto una serie di audizioni visto che - è stato già ricordato da altri colleghi -

Abbiamo svolto circa 70 audizioni, oltre ad aver raccolto molto materiale da parte di tutti coloro che volevano dire la propria rispetto a questo testo di legge. 70 audizioni sono tante e trovo francamente scandaloso - lo dico con piena coscienza - il fatto che una certa parte di questo emiciclo trovi inadeguato il numero delle audizioni

per cui sono state svolte 120 audizioni. Il mio Gruppo, la Lega, non ha detto di non voler fare 120 audizioni.

e mi auguro che lo sia solo per ora, perché anche quella è una tematica che non deve essere abbandonata e deve essere sostenuta. A noi, invece, cosa succede? Ricordo distintamente che, all'inizio della pseudo-discussione in Commissione sul disegno

così com'è. Sono notoriamente un *fan* del bicameralismo perfetto, perché credo che il confronto in più sedi possa portare a una norma più efficace e realmente pluralista.

perché credo sia un privilegio rappresentare il popolo e i cittadini e credo veramente in questa missione. Alcuni mesi fa, durante una seduta di Commissione - eravamo in sala Zuccari: lo ricordo molto bene - ho assistito a uno spettacolo sinceramente vergognoso,

veramente uno spettacolo indecoroso, tant'è vero che io, che prima avevo taciuto perché volevo ascoltare - mi hanno infatti insegnato che prima di contribuire, bisogna ascoltare le idee degli altri altri - in quella occasione ho preso la parola e ho manifestato tutto il mio disagio e, perdonatemi, anche il mio schifo, nell'assistere a come la funzione parlamentare possa scendere in basso. A tratti l'abbiamo visto anche nelle sedute

La discussione che si doveva intavolare non andava improntata sulla tutela di una serie di persone o di un'altra, ma dovevamo improntarla sul rispetto. Possiamo parlare di tutto, ma se non parliamo di rispetto per tutte le categorie, non andiamo a centrare l'obiettivo.

mente. Non voglio fare attacchi personali, assolutamente. Ieri la senatrice Maiorino ha detto che al centro ci devono essere le persone e che oggi non ci sono gli strumenti per tutelare le persone che

«Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All'umanità che ne scaturisce. A costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare… A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco». (Pier Paolo Pasolini).

questo è un caso in cui si dovrebbe parlare di dialogo tra sordi; ma in realtà è un dialogo tra un sordo e una parte dialogante. Qui c'è una parte politica che rifiuta di accogliere proposte emendative, sostenendo che il testo vada già bene così. Eppure in audizione sono state sollevate delle critiche. Penso ad esempio all'audizione del procuratore capo Domenico Airoma, il quale, sottolineando il suo intervento meramente tecnico, da operatore del diritto chiamato ad applicare le norme, ha detto, in buona sostanza, che alcune parti del provvedimento sono prive dei necessari requisiti di tipicità e tassatività della fattispecie incriminatrice; come a dire che l'area di ciò che è penalmente rilevante è incerta. Il testo contiene l'introduzione di un'aggravante speciale e su tale aggravante speciale noi abbiamo già detto di non avere particolari obiezioni, se non quelle relative eventualmente a una migliore formulazione del testo. Il

e corretto; l'idea che si possa commettere un reato perché magari mossi da odio verso una persona LGBT suscita riprovazione e repulsione. Ma il testo non si è fermato a questo; il testo ha cercato di fare assai di più. Mi riferisco a quella parte del testo dove viene introdotta una vera e propria nuova fattispecie incriminatrice, quella su cui ha concentrato la sua attenzione in audizione il procuratore (e non solo lui). L'ho citato perché il procuratore ha parlato da tecnico. La norma prevede la reclusione per chi istiga o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale

a quell'esercente di un pubblico esercizio che, fuori dalla sua discoteca, scrive: «Qui non entrano gli omosessuali». Certo, questo suscita indignazione, ma il problema è

il colore della pelle, la pigmentazione vale quanto la lunghezza dei capelli o il colore degli occhi, non vale nulla davanti alla legge

esiste geneticamente la differenza tra uomo e donna e questo non possiamo negarlo, tanto che addirittura le persone transessuali desiderano cambiare sesso, a riprova che c'è una differenza. Evviva quella differenza, dissero. Si crea un problema quando si tipizza una fattispecie incriminatrice che intende colpire la discriminazione per motivi di sesso, che possiamo forse anche punire; già esistono altre sanzioni per il pubblico esercente che impedisce l'ingresso nel locale agli omosessuali, ma - perché no? - anche ai meridionali o agli immigrati, per quanto possano essere regolari. Tuttavia diventa reato reato o quantomeno integra gli estremi materiali del reato il dar vita ad un'organizzazione che intende sostenere solo la genitorialità eterosessuale, perché anche questa diventa tecnicamente una discriminazione; tutti pensano che sia una discriminazione ragionevole, ma la norma non permette tale distinzione. Da questo punto di vista la norma è tecnicamente sbagliata perché basterà incriminare anche una sola volta una persona che intenderà distinguere sulla base delle sue convinzioni sociali e religiose, per intimidire tutti gli altri a manifestare la loro opinione. Questo non deve accadere, perché il diritto penale non serve a colpire un bersaglio sparando a pallettoni. Il diritto penale è una cosa seria, che richiede norme precise e puntuali, perché colpire anche un solo innocente in nome di un ideale che si ritiene giusto vuol dire essere dei giacobini e sappiamo per per quale ragione la storia ha consegnato questo nome a tristi ricordi. Devo dire che ieri - e lo dico con orgoglio e vanto - è stato un onore avere un colloquio con Franco Grillini, con cui ho discusso di questi problemi. Franco, che colgo l'occasione per salutare, mi ha detto di fare attenzione perché la norma che critico e in realtà è presente in tanti altri ordinamenti. Ha ragione, è vero. Sono andato a cercare, operando uno studio di diritto comparato, in quali altri ordinamenti c'è qualcosa di simile: ebbene, c'è una norma assai simile alla nostra, a quella di cui stiamo parlando, nell'ordinamento spagnolo, nel *codigo penal.* Non ve la leggo, ma è più o meno sovrapponibile a quella in discussione. Da qui l'estensore della norma ha preso il passaggio. Allora se c'è in Spagna va bene? No, perché per fortuna Internet non è solo il luogo dove ci insultiamo, alla faccia della tolleranza, su Facebook, ma è anche il luogo dove è possibile scaricare articoli scientifici. Se consultate Google Books o Google Scholar, troverete molti articoli in spagnolo che segnalano le gravi difficoltà interpretative che si accompagnano all'applicazione di questa norma. In Spagna stanno avendo gravi difficoltà a stabilire quale sia il discrimine tra la discriminazione lecita e quella illecita, tanto che nel 2019 si è resa necessaria una circolare della procura generale della Repubblica spagnola, volta a chiarire ai pubblici ministeri come applicare la disposizione. Queste incertezze durano ancora oggi, tanto che qualcuno ha proposto di abrogare la norma. Allora, se qualcuno prima di noi ci ha già provato e i risultati sono deludenti, se c'è in Spagna la preoccupazione che quella norma possa comprimere la libertà di manifestare le proprie opinioni, perché noi dobbiamo commettere lo stesso errore?

Dobbiamo stabilire se consentire a un collega come Simone Pillon di dire la sua. Simone Pillon, che molti di voi contrastano, va contrastato con le opinioni, non mettendogli il bavaglio, non impedendogli di parlare. Se volete contrastarlo, fatelo con le idee, fatelo con gli argomenti, fatelo con il ragionamento, ma non minacciando una sanzione penale. Nelle scuole bisogna insegnare la tolleranza. C'è un *lapsus* all'interno della norma: mentre la sanzione penale è volta a tutelare anche i disabili, vi siete dimenticati dei disabili nelle norme che invece intendono insegnare la tolleranza nelle scuole. Allora fatemi capire: va bene proteggere i disabili con la norma penale, ma poi agli studenti cosa insegniamo? Che esistono categorie più meritevoli di protezione, ancorché deboli, a scapito di altre? Non va bene. Nelle scuole dobbiamo insegnare ai ragazzi a essere dei buoni cittadini, a rispettarsi gli uni con gli altri e non si dà questo insegnamento se noi per primi rifiutiamo il dialogo e riteniamo che la controparte sia oggettivamente nel torto, a prescindere. Questo testo deve essere riformato, nel bene, a vantaggio di quelle categorie che vogliamo difendere. Non c'è l'infallibilità di una Camera a scapito dell'altra. Questo è un bicameralismo che serve proprio a correggere gli errori, a riflettere e a capire dove poter intervenire per consegnare all'ordinamento un testo chiaro e di facile applicazione.

non parla di adozioni e non parla di teoria *gender* o di altre situazioni che ho sentito nominare in quest'Aula; parla di una cosa molto semplice: come ampliare le fattispecie dei crimini di odio anche alle discriminazioni e agli atti di violenza compiuti in ragione del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere di una persona. Si chiede, quindi, di ampliare la norma e tra l'altro solo nella parte relativa all'istigazione alla violenza e non anche alla propaganda, come già per i crimini dovuti a motivi di razza, etnia, nazionalità e religione. Sul tema dell'omo-lesbo-bi-transfobia e di altre discriminazioni il nostro Paese ha sacche di arretratezza gravi e ciò non può essere negato o sminuito. Secondo Eurobarometro l'Italia, tra i Paesi avanzati, è tra quelli in cui la popolazione ha più difficoltà nell'accettare una società paritetica, al punto di ritenere, in gran numero, che gli omosessuali non debbano avere gli stessi diritti degli eterosessuali. È dunque una questione, questa, che non dovrebbe vederci schierati in opposte tifoserie, ma impegnati ad agire per mutare lo stato delle cose, ben consapevoli che i diritti e le libertà non sono affatto tutti uguali e che i diritti naturali, ovvero la libertà di esistere, essere, vivere e vivere appieno la propria esistenza, senza paura, vengono prima del fatto che si possa sentirsi liberi di esprimersi, al punto da minare l'altrui dignità. La libertà dalla paura è la prima delle libertà, perché, senza questa, tutte le altre non sono fruibili, sono libertà vuote. Quanto affermo era ben chiaro a John Locke quando disse che vi era un limite di tolleranza verso l'intolleranza e che, appunto, la libertà non è priva di confini. Non siamo infatti liberi di uccidere né di rubare; non siamo parimenti liberi, dunque, di minare la serenità e la sicurezza dell'esistenza di un altro essere umano in virtù di un pregiudizio sulla sua natura. Tutto questo è chiaro anche alla nostra Carta costituzionale, che enuncia nei suoi primi 12 articoli i principi fondamentali della nostra Repubblica e che agli articoli 2 e 3 ci parla, appunto, dei diritti inviolabili dell'uomo, quali la pari dignità sociale senza alcuna distinzione, al punto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 21 circa la libertà di espressione, in ogni modo niente affatto minato da questa legge, come già chiarito da numerosi costituzionalisti, seppur importante, viene dopo, molto dopo gli articoli 2 e 3. Data l'importanza delle tematiche in oggetto, dunque, sarebbe stato un bel segnale avere maggiore condivisione da un lato e più mediazione dall'altro. Credo che abbia sbagliato chi, in una fase iniziale, quando il disegno di legge era alla Camera, ha scelto di tenersi fuori dal dibattito, talvolta usando anche atteggiamenti pretestuosi o argomentazioni palesemente inesatte; ma allo stesso modo credo oggi che sbagli chi si ostina in posizioni di chiusura a un ulteriore confronto, delegittimandone le finalità. Penso che si debba provare fino all'ultimo perché, comunque la si voglia mettere, un ultimo miglio possibile per un tentativo di incontro c'è ancora. Non sto dicendo che porterà a un risultato - questo non posso saperlo - ma so che è necessario provarci se davvero qui teniamo tutti ai diritti e non alle bandiere. Rivendico in Forza Italia un atteggiamento costruttivo, anche nel lavoro in Commissione già ai tempi della Camera; ma all'epoca, l'eccessiva polarizzazione delle parti, per cui non vi era stata l'apertura al dialogo che c'è stata qui, ha portato al lavoro che non è uscito bene: prova ne è quell'articolo 4 da noi voluto che forse è, secondo il mio parere, quello più critico della norma, più ridondante, più lacunoso e più insidioso. In questo ramo del Parlamento è cambiato qualcosa e finalmente sento anche meno nominare le statistiche a supporto di chi sostiene che si sta parlando di un non problema per il basso numero di casi di violenza specifica denunciati. Si sta iniziando a comprendere che tali dati non sono corretti, perché altri dati e statistiche ci dicono che, purtroppo, invece, il nostro Paese è messo molto male a livello di tolleranza e rispetto, come ho già detto.

L'*under-reporting* è la difficoltà della vittima nel denunciare l'aggressione subita per quello che è, per paura, vergogna e per tanti altri motivi, mentre l'*under-recording* risponde alle difficoltà, per gli organi di Polizia, di registrare il dato correttamente, anche qui per vari fattori, non ultimo perché manca la norma specifica in cui catalogarli. Quindi, è proprio necessario occuparsi di ampliare il perimetro dei crimini di odio, colmando un vuoto normativo. I crimini di odio sono crimini specifici; chi ne è vittima, lo è per quello che rappresenta con la sua identità di essere umano, non è una vittima per una casualità futile. Il motivo è legato all'essenza, alla dignità, alla libertà di esistere di quell'individuo e alla comunità che rappresenta. Il motivo è sostanza, è significante e infine, se si accetta che si sia dedicato il 604*-bis* del codice penale per motivi che esulano dalla natura dell'individuo, suppongo che lo si possa accettare anche per questo. questo. Va detto, poi, che alla vittima di umiliazione e discriminazione importa il giusto di sapere che vi sarà una pena più severa; ciò che è davvero importante è altro, ovvero vivere in una società adulta, matura, educata al rispetto. La società civile è a maggioranza consapevole; gli italiani si dicono favorevoli a una legge di questo genere (...) scusate...

Va detto che alla vittima di umiliazione importa il giusto, quello che importa è una società educata al rispetto. La società civile è a maggioranza pronta e consapevole. Gli italiani infatti si dicono favorevoli ad una legge di questo genere, addirittura anche a questa, così com'è, pur con tutte le criticità, alcune oggettive, e i timori che sono stati trasmessi loro. Fra questi italiani favorevoli, dato che i numeri non sono opinioni, ci sono anche elettori di centro destra. Per il mio partito si parla del 48 per cento di favorevoli; saranno meno o di più il punto non è questo. Il punto per me è rispondere a chi voglia ritenere che una posizione come la mia non sia propria di un certo elettorato, perché invece lo è. Certo, ripeto, arrivare a un percorso più ampio e condiviso, limando alcune vaghezze, senza con ciò stravolgere l'impianto normativo, sarebbe auspicabile e l'atteggiamento di chiusura e solo forzatura non fa bene né ai diritti, né alla democrazia. So però che giunti a questo punto sarebbe grande la sconfitta di vedere ancora una volta morire un disegno di legge per il quale, in venticinque anni, tutte le volte che è stato tentato un *iter* legislativo, non è stato poi terminato ed è stato affossato in uno dei due rami del Parlamento. anni che una comunità di persone è costretta a sentirsi figlia di uno Stato minore; venticinque anni in cui l'Italia indietreggia rispetto a posizioni di civiltà presenti negli altri Paesi a noi fratelli per cultura e livello democratico, dove leggi come queste sono state votate da Governi di tutti i colori politici. Quando capì Quando capì di me, mia madre mi disse «ho paura per te»; tutti i genitori hanno paura per i propri figli, per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino, ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è. A voi tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari, quelli di oggi e quelli di domani, e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri e poter dire loro «io, nel mio piccolo, ti ho protetto dalla paura». Ringrazio la mia capogruppo Anna Maria Bernini, i miei colleghi senatori e il mio partito Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre dimostrato. Grazie, senatrice Masini, l'abbiamo ascoltata con molta attenzione. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo il disegno di legge Zan ha l'obiettivo di proteggere tutti, la comunità LGBT, le donne, gli uomini, i disabili, dai cosiddetti reati dell'odio, cioè l'istigazione a commettere atti violenti o discriminatori nei loro confronti. Il disegno di legge di cui oggi discutiamo, già approvato alla Camera dei deputati, si compone di diversi articoli attraverso i quali si modificano i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale per aggiungere alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, anche gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. L'espressione orientamento sessuale è già utilizzata nella legislazione italiana, ad esempio, nel codice della *privacy*, il cui articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. L'espressione identità di genere si ritrova, ad esempio, nell'ordinamento penitenziario all'articolo 1, dove impone di improntare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità senza discriminazioni in ordine, tra l'altro, al sesso, all'identità di genere e all'orientamento sessuale. legge, che ci auguriamo concluda il suo corso con l'approvazione, interviene solo contro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione e di violenza. Siamo l'ultimo Paese tra i fondatori dell'Unione europea a non avere una normativa penale in tal senso. C'è una forte necessità di tutelare le vittime e di prevenire la violenza di ogni tipo, sia fisica che verbale, e per comprendere la necessità e l'urgenza di una giusta legge contro la misoginia e l'omotransfobia è sufficiente guardarsi intorno, aprire le pagine di un giornale e semplicemente parlare con le vittime delle discriminazioni, le vittime dell'odio

Per questo è una legge necessaria e urgente, perché l'Italia ha bisogno di rafforzare la cultura dell'uguaglianza e del rispetto per l'altro e questo può avvenire punendo l'odio e la violenza, promuovendo concrete azioni sul piano culturale e sociale per il sostegno delle vittime, per spiegare e far capire che la diversità non deve far paura, ma è una peculiarità della natura, com'è la biodiversità, e come tale deve essere valutata o - io direi - rivalutata. Ed è esattamente questo che fa il disegno di legge Zan: prevenire, contrastare, sostenere, sensibilizzare, creare unione e non divisione. I fatti di cronaca denunciati da numerosi quotidiani nazionali e locali hanno segnalato l'esponenziale aumento, sia nel numero che nella gravità, di atti di violenza, azioni legate a discriminazioni, per motivi di orientamento sessuale e di identità di genere orientati a colpire il diverso, a colpire i disabili. La legge prevede anche un recupero di chi commette il reato tramite vari percorsi all'interno di organizzazioni di volontariato. In questo senso la sanzione sarà rieducativa, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione. Inoltre, si mettono in campo iniziative di formazione nelle scuole per combattere il bullismo omotransfobico e di ogni altra forma. E qui torno ai disabili: certo, in questi giorni fa molta più scena parlare delle diversità collegate al sesso, ma semplicemente perché la nostra società è abituata a trattare ciò è di forte impatto, ma pochi hanno posto la loro attenzione sui disabili, che sono fortunatamente previsti dal disegno di legge, i cosiddetti portatori di *handicap*. Certo fanno meno scalpore, perché continuano a restare nell'ombra, ma l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità le riconosce per la prima volta in modo esplicito come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Il principio sancisce che essere una persona disabile non è meglio o peggio rispetto a non esserlo e che non sono le caratteristiche di un individuo a definirlo svantaggiato, ma il contesto in cui è inserito. In altre parole, la disabilità è il risultato dell'interazione tra condizioni individuali, definite fuori dalla norma, e una società non preparata ad accoglierle. Non a caso in inglese le persone con disabilità vengono dette «disabilitate», rese non abili dal contesto, costruito a misura di cittadini normodotati. Le discriminazioni contro i disabili ci sono: si chiamano abilismo, sono manifestazioni di violenza abilista, le aggressioni fisiche o verbali, come «sei un handicappato» o «sei un Down». Notizie continue di cronaca denunciano episodi di violenza vera e propria, come quelle avvenute in una struttura residenziale per ospiti disabili a Palermo, o di aggressioni come quella subita da una ragazzina con disabilità, picchiata da un gruppo di coetanei a Roma, o ancora in casi di maltrattamento di persone disabili da parte delle loro famiglie. Esiste poi una forma di abilismo più subdola, cioè la tendenza a definire le persone unicamente in base alla loro disabilità, riferendole in modo stereotipato e connotando la loro diversità con un senso di inferiorità. essere una donna disabile è più stigmatizzante di essere una donna abile o un uomo disabile; essere una donna lesbica o trans con disabilità ha un impatto ancora più grande. L'essere donna è condizionato dall'essere una persona disabile o viceversa, come anche essere lesbica o trans condiziona il proprio modo di vivere la femminilità e la disabilità. Dove voglio arrivare? che l'essere donna, trans, disabile ed omosessuale non sono blocchi monolitici, ma si influenzano a vicenda: le persone LGBT con disabilità sono vittime di discriminazioni multiple, esattamente come le donne disabili, perché le discriminazioni non si sommano, ma si moltiplicano. Non posso dimenticare i disabili. Non sapete cosa significhi quando tua figlia torna a casa e ti dice: «Mi hanno detto che sono diversa. Non sono come loro e non posso quindi giocare con loro»; oppure quando torna con la felpa tutta disegnata con scritte poco piacevoli o si sono inventati un gioco per beffarsi di lei,

Quello che cerco di dirvi è che la situazione è delicata. Confido in uno sforzo di coesione nella maggioranza: è il momento di vincere le paure, di avere il coraggio di cambiare in meglio e di andare oltre, per unire con un filo la rete della vita. Questo disegno di legge non danneggia nessuno e non toglie diritti; semmai, aggiunge un tassello in più al mosaico dell'uguaglianza nel nostro Paese. Noi del MoVimento 5 Stelle supportiamo questo disegno di legge, perché da sempre il MoVimento è per la difesa dei diritti di tutti e soprattutto di coloro che spesso sono dimenticati, perché in questo unico Pianeta che abbiamo siamo una sola e unica comunità.

il dibattito che stiamo affrontando oggi non è per nulla scontato e neppure secondario, come qualcuno vuole strumentalmente farci credere. Siamo in Aula ad affrontare una discussione in merito a un disegno di legge che altro non è che un bavaglio imposto dalla dittatura del pensiero unico che, usando la scusa delle discriminazioni, peraltro già punite dall'attuale ordinamento, con relative aggravanti, tenta in realtà di eliminare ogni possibile voce di dissenso. Il disegno di legge Zan è ideologico, profondamente sbagliato e antidemocratico. La verità è che, dietro a molti esponenti del politicamente corretto che oggi si battono per questa proposta, si celano in realtà colossi della finanza e del *marketing*, che promuovono uno stile di vita consumistico, intento ad annientare ogni forma di identità e differenza, dal genere al pensiero dissidente. Il piano è chiaramente quello di creare un esercito di burattini, che, mercificando le loro vite e facendosi profilare in tutto e per tutto, vadano a formare l'archetipo del perfetto consumatore, annullando ogni scelta personale. *(Applausi)*. vorrebbe vivere in una società che neghi le figure del padre e della madre per quelle del genitore 1 e del genitore 2: non più maschio e femmina, un essere indeterminato e autodeterminato, con il paradosso di non fermarsi al genere umano. Se così fosse, cosa potremmo fare, se un domani qualcuno dovesse sentirsi di appartenere al genere animale oppure di provenire da un altro pianeta? L'eccesso di libertà provoca inevitabilmente un annullamento della verità, portando caos normativo e annacquando i giusti provvedimenti che già esistono contro le discriminazioni. Siamo convinti, cari colleghi, che in politica le giuste e doverose rivendicazioni dei diritti debbano seguire un binario legislativo ben preciso, altrimenti rischiamo un cortocircuito, come nel caso del Zan, di cui oggi stiamo discutendo. Ad oggi, esiste già un numero potenzialmente illimitato di generi: ad esempio, il famoso *social network* Facebook, nelle fasi di iscrizione, ne censisce già diversi, ma questi come possono essere determinati e identificati, se il genere è una scelta arbitraria e non biologica? Come porre limiti per legiferare e certificare l'appartenenza, più o meno duratura nel tempo, a un certo genere? Se una persona ogni giorno ne sceglie uno diverso, come adottare misure di sostegno a una determinata categoria, come nel caso delle quote rosa, del femminicidio, del lavoro delle diverse categorie, delle discipline sportive e dei regimi carcerari? Affermiamo sempre più spesso il valore della parità di genere e dell'esserci dimenticati delle differenze, anzi delle bellissime differenze di genere che la natura ha creato tra uomo e donna. Se non ci sono differenze, vorrà dire che domani tirare un pugno in faccia a un uomo o a una donna avrà lo stesso impatto sociale? I maltrattamenti sulle donne e sugli altri generi autodeterminanti saranno parimenti sanzionati? Capite, colleghe e colleghi, che, senza differenze, né direzione, non ci sarebbero più tutele per le categorie più fragili? Questa è una vera e propria discriminazione al contrario. disegno di legge Zan solo come una proposta per aggiungere all'elenco delle categorie particolarmente protette dalla legge Mancino anche quelle dei discriminati per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere è estremamente fuorviante. Chi non sarebbe d'accordo con questo? Discriminare qualcuno per futili motivi, perché si veste in un certo modo o è omosessuale, è assolutamente folle e va punito severamente, ma siamo davvero sicuri che allungare l'elenco di queste categorie non costituisca di per sé un discrimine nei confronti delle altre? I senzatetto, le persone sovrappeso, quelle con disturbi psichici o semplicemente con una corporatura più fragile sono forse più discriminabili? No, cari amici: la verità è che bisogna riconoscere che già adesso la legge punisce severamente ogni forma di discriminazione, comprendendo già

A riprova del fatto che il disegno di legge Zan è orientato, più che a combattere le discriminazioni, ad affermare una nuova ideologia, basterebbe osservare con attenzione le stesse proposte di legge che l'onorevole Zan e altri hanno presentato in passato, cui tutti i riferimenti all'identità di genere, all'indottrinamento scolastico e agli altri punti controversi non erano nemmeno considerati (come nel disegno di legge del 2013,

Se fosse stato solo un disegno di legge contro le discriminazioni, probabilmente l'avremmo votato tutti all'unanimità, ma la verità è che il disegno è molto differente e subdolo. Non solo, ma ad oggi - dobbiamo ricordarlo - non risulta esserci in Italia un'emergenza legata al problema dell'omotransfobia, cioè una diffusione allarmante di violenze o discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, necessari ulteriori interventi del legislatore. Benché il nostro Paese venga percepito - anzi, venga fatto percepire - da qualcuno come omofobo, i dati non supportano questa suggestione mediatica. Union Agency for Fundamental Rights (FRA) dell'Unione europea hanno rivelato, sia nel 2014, sia nel 2020, che l'Italia è tra i Paesi più sicuri d'Europa per quanto riguarda concreti episodi di violenza, minaccia e discriminazione.

e di sostenere la propria contrarietà a una minoranza che continua ad arrogarsi il diritto di imporre una propria visione. Tuttavia, noi di Fratelli d'Italia, per difendere i principi e i valori che hanno forgiato la nostra cultura millenaria, continueremo la nostra battaglia di libertà, senza odio e senza alcuna discriminazione. Lo faremo consapevoli di andare controcorrente, con l'unico scopo di non permettere l'annientamento della nostra civiltà, condannata a soccombere contro un male che la sta annullando in modo irreparabile.

Signor Presidente, inizialmente non avevo molta intenzione di intervenire sul tema, nonostante a me piaccia molto il dibattito e, anzi, qualcuno giustamente mi faccia notare che parlo anche troppo.

non possiamo sicuramente andarci a impantanare in un tema divisivo, a maggior ragione perché, tra l'altro, sempre il Presidente del Consiglio, sostenuto peraltro da una larga maggioranza, aveva cortesemente chiesto di evitarne. *(Applausi)*. Cosa facciamo, dunque? Naturalmente, mi assumo la mia quota di responsabilità, perché ho sottovalutato la questione, lo ammetto.

improvvisamente in Aula, senza un'analisi in Commissione. Alla fine, probabilmente, le famose mediazioni avremmo potuto trovarle lì. Ne abbiamo trovate tante,

Penso che ci sia un punto fondamentale. Pongo la domanda a me stessa e la rivolgo a tutti voi. Secondo voi, quando si andrà a votare, nel 2022 o nel 2023, 2023, le forze politiche riceveranno un giudizio dai cittadini sulla base di questa contrapposizione, che durerà tre o quattro giorni, o di quanto e come abbiamo sostenuto l'azione di un Governo che

anche perché lo stare insieme, come vediamo tutti i giorni, è una questione che pesa. Non riesco a capire per quale motivo si debba portare il peso, da una parte, e non si debbano raccogliere i risultati, dall'altra, quando poi abbiamo un Governo che i risultati li porta a casa e parla poco. Quindi, dovremmo parlare noi; dovrebbero essere le forze politiche a spiegare ai cittadini cosa si sta facendo di buono. Invece, stiamo una settimana a discutere di questo,

e ha parlato chiaramente di una disfatta collettiva. Non possiamo essere distonici completamente rispetto a ciò che fa il Governo. Potremo scivolare in qualche bandierina, ma non aver fatto una divisione di questo genere, secondo me, è distonico e sbagliato, perché c'erano mille modi per affrontare questo disegno di legge.

questo. Abbiamo problemi e lo sappiamo benissimo, perché se n'è discusso anche alla Camera, e le questioni fondamentali sono relative al concetto di istigazione. Non lo sto a ripetere, in quanto l'hanno spiegato tanti colleghi molto meglio di me. molto meglio di me. Rischiamo di avere un ordinamento in cui nella pratica il confine sottile tra la libertà di pensiero e l'istigazione può diventare deflagrante.

Credo che sia giusto e che sia anche il tempo che ci concentriamo su quelle, perché, secondo me, prima della pausa estiva, dobbiamo mettere alcuni punti sulle riforme che riguardano il settore della giustizia. Lo dobbiamo fare nella nostra Commissione, con tutti i pareri annessi e connessi, che attengono naturalmente alla Commissione bilancio. Concludo dicendo

No). Credo che sia una ipocrisia, perché chi vuole che effettivamente un disabile non sia discriminato deve avere il coraggio - che, non so perché, non riusciamo ad avere - di cambiare, tanto per cominciare, la legge n. 68 del 1999, perché il disabile è umiliato e discriminato nel momento in cui cerca un lavoro, che - lo sappiamo benissimo - le aziende non gli danno, perché preferiscono pagare la multa. *(Applausi)*. Questo è molto più scandaloso,

innalzate solo a seguito di una sentenza della Corte costituzionale. *(Applausi)*. Rispetto le posizioni di tutti e sto in Forza Italia per questo, per

è da mesi che siamo chiusi qui in Senato per fare questa discussione e ogni tanto mi sembra che veramente viviate su Marte. Se aprite i giornali anche voi,

le pene per chi discrimina in base all'orientamento sessuale e alle proprie vocazioni. Su questo siamo d'accordo. Se l'obiettivo comune è quello, ritengo che in quindici-venti giorni o in un mese

identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Cosa significa? Dobbiamo spiegarlo. Mettiamoci d'accordo sull'aumentare le pene a chi discrimina. Andiamo a leggere ad esempio l'articolo 4, che secondo me è veramente il più preoccupante di tutti.

o aiutare? Qual è il vostro obiettivo? Fermiamoci. Se l'obiettivo comune è dare una pena maggiore a chi discrimina, facciamolo. Perché dovete introdurre tutti questi tasselli, che vanno poi

fermiamoci, ragioniamoci e approviamo l'aumento delle pene per chi discrimina, ma tutto il resto togliamolo. Su questo la Lega c'è, noi ci siamo; facciamo di questa legge qualcosa di buon senso

nelle scuole, al lavoro, nella vita di tutti i giorni e in politica. Per noi, senza fare del vittimismo che sicuramente non ci appartiene, a volte è stato difficile anche solo esprimere le nostre idee. Abbiamo sofferto una discriminazione che è arrivata fino alla violenza,

chi è discriminato a sentirsi meno solo, più accettato e più integrato nella società, perché chiunque ha il diritto di essere felice e di vivere compiutamente la propria esistenza.

legge dire che c'è un complotto delle destre oscurantiste per oscurare tale progetto di civiltà.

di disagio vero, intimamente rilevante, che pure ci sono e delle quali dobbiamo occuparci. La verità è che questo movimento trae la sua linfa vitale dalle multinazionali, da chi gestisce i network,* dalle grandi produzioni televisive e dai grandi centri di poteri finanziario. Tutto questo meccanismo è allineato nella promozione del movimento LGBT.

per un bambino sia opportuno avere un padre e una madre di sesso diverso, l'ordine dei campioni del globalismo e del progressismo più estremista (gli *influencer,* i cantanti, i calciatori e tutto lo *star system*: conosciamo bene lo schema, perché è già "accaduto" negli Stati Uniti d'America) è quello di ghettizzare tutti coloro che la pensano in maniera diversa, a cominciare dall'Est della nostra Europa: i barbari di Orbàn e quegli Stati canaglia che hanno soltanto una visione più tradizionalista della vita sono da punire, però nessuno dice una parola

quando va bene, viene vista come una malattia, e, quando va male, viene punita con la pena di morte. *(Applausi)*. Invece di parlare di Orbàn, vedete chi state facendo entrare in questo momento dalle nostre frontiere.

Dove sono le multinazionali del pensiero unico? *(Applausi)*. Dove sono le sirene del buon senso e della civiltà, nonché le bandiere arcobaleno nelle scuole? Dove sono? Prima vengono i soldi, poi è chiaro che ci stanno i diritti. Prima il dio denaro.

questa proposta è sotto gli occhi di tutti. Pretendono di pianificare una società in cui non esistono principi non negoziabili, si allargano diritti si distruggono, si disintegrano e si stravolgono le identità, senza pensare che, sgretolando le radici, si fa un danno a tutte le persone, soprattutto a quelle più deboli. Il vero rischio, com'è stato già detto, è che questo megaesperimento sociale, che è alla base dei fenomeni che gestiscono come grandi burattinai questo mondo, in realtà, dietro una finta promozione dell'amore, nasconda una propaganda di odio, di violenza e, quello sì, di vera discriminazione.

ci sono momenti nella storia di un Paese che segnano passaggi epocali. Sono momenti importanti, in cui si comincia a costruire il percorso che porterà la società

a renderci più democratici e civili. Si tratta di momenti così importanti che chi ne è protagonista in prima persona dovrebbe sentire forte la responsabilità che porta, ponendosi nella migliore disposizione rispetto all'apertura di dialogo, al confronto e alla mediazione, per giungere a un risultato di partenza condiviso. È il caso del momento segnato dalla discussione del disegno di legge recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Partiamo da un presupposto essenziale, innanzitutto, quello del profilo procedurale e poi di merito. Siamo il Senato della Repubblica, uno dei due rami del Parlamento, con pari poteri, doveri e dignità: va bene che noi siamo modesti e generosi, ma perché tanto clamore e tanta fretta di chiudere un provvedimento così delicato e volerlo lasciare così com'è, quando alla Camera ci è rimasto per più di un anno? Sono convinta che tutto il *can-can* mediatico e *social*, l'ideologizzazione selvaggia, l'intransigenza e il muro alzato contro ogni mediazione, per poter piantare una bandierina partitica, siano quanto di più sbagliato per affrontare un tema come quello dei diritti LGBTQ e dell'istigazione alla discriminazione e all'odio, che dovrebbe essere, invece, trattato in maniera seria, alta, trasversale e profonda, trattandosi di una materia di civiltà, che dovrebbe unire e renderci più forti e non dividere. Il disegno di legge in esame, nascendo a tutela dei diritti e del rispetto della persona e della libertà individuale, proprio da questi principi imprescindibili dovrebbe essere retto. un provvedimento che non avrebbe dovuto neanche avere un cognome e che dovrebbe segnare una svolta nel sistema culturale e sociale di una Nazione, che dovrebbe trovare un punto di incontro e non punti divisivi, che lascerebbero aperto uno scontro che non dovrebbe mai più esistere. Invece, il padre del disegno di legge cosa afferma? Cosa dice? Dice che non si media sulla pelle delle persone. Cosa vorrebbe sottendere quest'affermazione? Che deve semplicemente vincere il più forte? Che ce la dobbiamo giocare a braccio di ferro e chi butta il braccio dell'altro sul tavolino vince? Che ci dovremmo dividere in buoni e cattivi? Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo essere semplicemente spettatori. Le poltrone di quest'Aula non sono quelle di un cinema e noi non siamo, non vogliamo e non possiamo essere spettatori passivi. Siamo i rappresentanti del popolo, di tutto il popolo, e una legge equa e giusta deve trovare un punto di incontro e non di scontro, non creare spaccature sociali. Qui rischiamo di snaturare il ruolo altissimo del Parlamento, e sottolineo del Parlamento, non di un *social* o di un dibattito al bar. Una legge di civiltà, di evoluzione culturale, dovrebbe essere una legge di pacificazione, non di divisione; dovrebbe trovare un punto ideale di mediazione per diventare davvero un momento di evoluzione e non di involuzione. Non dovrebbe, nel corso della discussione, avere fuori dal palazzo la polizia per paura di scontri; non è possibile che una legge contro l'odio generi odio a tal punto da aver creato due tifoserie contrapposte. Questo non è buono. È la base. Senza condivisione e pacificazione non avrà vinto nessuno, e qui non si tratta di far vincere una parte o l'altra, ma di far vincere la libertà, i diritti, il rispetto. Per Forza Italia il rispetto della dignità della persona umana, la tutela delle libertà individuali, ma anche la tutela del diritto pubblico vengono sopra tutto, ed è per questo che il nostro approccio è stato, è e continuerà a essere sempre molto serio. Non perdiamo questa importantissima possibilità di fare un grande passo avanti sociale e culturale. Non rischiamo - per il desiderio di taluni - di mettere una bandierina dimostrando integralismo intollerante, di gettare via tutto, di essere più contenti nel dire «è colpa loro se abbiamo perso» piuttosto che dire che abbiamo vinto tutti. Se ancora il bicameralismo perfetto regge il nostro potere legislativo non dobbiamo averne paura. È evidente - lo ripeto - che la politica è mediazione, come è evidente che questo Parlamento rappresenta tutti, ogni singolo cittadino che è entrato nell'urna di un Paese democratico e ci ha affidato la grande responsabilità di essere rappresentato. Ricordo quando in quest'Aula, proprio qua, da questo stesso banco, nella XVI legislatura fui relatrice di un'altra legge di civiltà, quella sulla equiparazione dei figli, per eliminare l'odiosa aggettivazione naturale e legittimo all'interno del codice civile, quindi le discriminazioni conseguenti; quella che io rinominai la legge Filumena Marturano: i figli sono figli. Anche allora si accese un dibattito molto serrato, ci furono veri e propri scontri, ma ce la facemmo, e in Senato, con grande orgoglio, la legge passò all'unanimità, perché alla fine ci sedemmo tutti insieme e appianammo le divergenze trovando i punti ideali di mediazione a tutela del nostro bene più prezioso, i figli. Oggi il punto di mediazione va trovato a tutela del bene supremo, la libertà di ognuno, peraltro garantita dall'articolo 21 della Costituzione, per arrivare a imparare a crescere nelle differenze, rispettando ogni persona in quanto persona. Fermiamoci per un attimo a pensare che il risultato delle prove Invalsi - oggi è su tutti i giornali - ha dato un esito, a mio avviso, da insegnante, da madre, da parlamentare, terribile, inquietante. I nostri ragazzi delle superiori sono fermi al livello delle medie. Su questo dovremmo correre ai ripari, altrimenti non avremo giovani in grado di sviluppare la propria coscienza critica per compiere le scelte migliori e per sviluppare le corrette sensibilità,

È un altro discorso, ma si inserisce serenamente in questo che stiamo trattando. Quindi, rispetto e tutela della dignità della persona umana senza distinzione alcuna vuol dire tutela e rispetto di ogni persona, quindi, anche di chi chiede di trovare un punto di incontro che consenta di licenziare questa legge facendo svolgere al Parlamento, la più importante istituzione della rappresentanza popolare, la sua funzione essenziale: esprimere la prerogativa più alta per garantire che il pensiero di ognuno trovi casa nella composizione di una legge. Non costringete questo Parlamento a un voto politico rispetto all'arroganza di un *leader* che lancia un *Diktat* senza se e senza ma e che essendo *leader* di una sola parte - il Partito Democratico nella fattispecie - costringerebbe gli altri a sentirsi condizionati in una scelta. Sono certa che anche all'interno del Partito Democratico ci sono, giustamente, sfumature di pensiero diverse tra loro che se fossi un *leader* di partito, tenderei a rispettare per non rischiare poi sorprese al momento del voto. questa legge più armoniosa in quanto legge di civiltà e di rispetto, più rispettosa dei *sentiment* dei vari movimenti di opinione. Anche l'opinione pubblica è spaccata e noi dobbiamo essere i garanti di un provvedimento che venga accolto nel migliore dei modi da tutti e che non diventi paradossalmente strumento di divisione e di scontro. Qui si parrà la *nobilitate* del Parlamento, qui si parrà la nostra capacità, la nostra serietà, la nostra volontà di voler davvero licenziare una legge fatta bene per tutti, come deve essere una buona legge. È in un momento come questo, su una legge divisiva non nel suo nucleo sostanziale, ma in sfumature molto delicate, che noi dovremmo dimostrare di meritarci il ruolo che ci hanno affidato i cittadini, riuscendo a fare quello che si dovrebbe fare su ogni provvedimento: trovare la sintesi ideale. Irrigidirsi sulle posizioni, parlare parlare di punti non negoziabili servirà solamente ad allargare sempre di più il divario politico e questa è l'ultima cosa utile per un provvedimento che gira una pagina della storia italiana.

Un perimetro pericoloso tra pensiero libero e offesa, che non ha una delimitazione chiara, lasciando ampio spazio alla discrezionalità di una terza figura; chi decide cosa è idoneo? Questo va specificato. Non stiamo parlando di amore, di sentimento, che non mettiamo in dubbio, ma del codice penale e quindi dobbiamo essere chiari. Serve certezza Serve certezza nella norma, c'è poco da fare. Non possiamo lasciare allo sbaraglio i cittadini senza una norma chiara. La libertà di opinione non può mai essere compressa, mai, e per questo ci batteremo in tutte le sedi, ovviamente sempre che essa sia canalizzata all'interno del rispetto culturale e della cultura stessa in quanto termine importante. È questo che mi fa riflettere, non accettare e rigettare l'appello della Lega al dialogo è un atto ideologico incomprensibile; trincerarsi dietro una posizione non condivisa da tutti è una dimostrazione di debolezza politica. Avete delle idee deboli e lo stiamo dimostrando tutti i giorni con i nostri interventi, articolandoli in nome della Costituzione italiana. È una debolezza che rischia di dare vita ad una nuova inquisizione, una moderna caccia alle streghe nei confronti di chi giustamente è convinto che la famiglia è composta da mamma e papà. Io stesso ho subito un linciaggio *social* per un *post* nel quale rivendicavo il ruolo dei genitori biologici, un linciaggio mediatico. Per questo esprimo solidarietà ai senatori Pillon, Ostellari e a tutti i miei colleghi che sono stati veramente linciati sui *social* perché hanno espresso la loro opinione libera: uomini coraggiosi, che vanno contro il pensiero unico. E con forza, appunto, voglio gridare: le idee non si processano, un modello di vita non si processa, un credo religioso non si processa. Vogliamo parlare dell'articolo 7, che istituisce percorsi all'interno della scuola? È un articolo molto confuso: non si specifica chi è tenuto ad organizzare questi corsi sull'omofobia e soprattutto con quali competenze. Parliamo di cultura *gender*? Se così fosse, mai e poi mai ci troverete d'accordo. Libertà per i ragazzi italiani e le ragazze italiane di crescere come credono, senza essere influenzati. Il pensiero unico non può essere l'unico dogma imperante; la diversità delle idee è il sale della democrazia.

la loro libertà a disposizione di tutti, perché da domani - ma sono convinto che non accadrà - potremmo essere meno liberi. È per questo che credo che ognuno sia libero di vivere la propria sessualità come meglio crede, ma ciò non autorizza nessuno né a limitare le libertà altrui, né a influenzare la crescita dei ragazzi. Sarebbe bello vedere tanta enfasi anche davanti agli innumerevoli crimini subiti dai cristiani nel mondo. ultimo caso (in molti, troppi, fanno finta di saperne poco o nulla, girano la testa): sapete che una giovane italo-marocchina di ventitré anni è stata arrestata in Marocco

sentimentalismo, leggendo i messaggi che mi arrivano. Prima erano tutti commossi e attenti ai messaggi che arrivano di gente che si sente discriminata, i quali hanno la nostra solidarietà, ma io vi leggo i messaggi che mi arrivano anche da altra gente che merita grande solidarietà dalla politica: i lavoratori. sinistra, infatti, ormai ha abbandonato la classe operaia per diventare serva delle *lobby*, anche delle *lobby* ricchissime che non hanno sicuramente né problemi economici, né di diritti. Ecco, i messaggi che mi sono arrivati: «Il fondo volo non è arrivato; a fine mese non riusciamo a fare la spesa. Però qui ce ne freghiamo, dobbiamo parlare di altro,

Lancio un messaggio all'intelligenza di sinistra, soprattutto a quelle persone che in questi giorni, credendosi di essere elevate sia sotto l'aspetto culturale che sociale, ci stanno criticando: noi non abbiamo paura e per difendere un'idea, per difendere la verità e per difendere la libertà siamo pronti anche alla galera. Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, vorrei innanzitutto fare alcune considerazioni sul metodo seguito. Siamo abituati, come Senato e come ramo del Parlamento, a ricevere disegni di legge già confezionati, pronti da approvare e di iniziativa governativa, che riguardano misure urgenti contenute in decreti-legge e che spesso riguardano temi economici o scadenze che vengono prorogate. Talvolta, e non di rado, ci è capitato anche di farlo attraverso voti di fiducia. parlamentare giunto dalla Camera dei deputati che non ha nessuna data oltre la quale il testo non sarebbe più valido. Eppure ci viene presentato come inemendabile, quindi come immodificabile, e l'unica testimonianza che ci viene concessa è quella di un intervento nell'Aula del Senato. Peraltro, questo testo ci viene esibito come il frutto della mediazione di tutte le forze alla Camera, e viene detto a noi moderati liberali di Forza Italia che il contributo dei nostri deputati è stato determinante per scrivere il testo ora in esame. È stato determinante il contributo di tutti, ma il nostro apporto di senatori non è richiesto: non possiamo proporre o approvare modifiche altrimenti si snatura la *ratio* del testo, frutto - si dice - di un equilibrio delicato. Ma il contenuto del disegno di legge Zan ha fatto manifestare forti preoccupazioni da parte del mondo intellettuale e dell'università, oltre che del mondo cattolico. Quindi non è, come qualcuno vuol far credere, che da una parte ci sono i rozzi e gli insensibili e dall'altra coloro che si prendono cura dei soggetti più deboli. La preoccupazione del mondo cattolico e accademico sta proprio nel fatto che si vogliono cristallizzare definizioni non chiare in norme giuridiche, alcune delle quali aventi carattere penale. scrivendole in forma normativa, a trasformare in dogmi delle definizioni che sono ancora oggetto di dibattito scientifico, ma che potrebbero cambiare, fino ad annullarlo, anche il concetto tradizionale della famiglia. si prova, dunque, attraverso l'introduzione di questi dogmi, a limitare la libertà di manifestazione del pensiero che - lo ricordo - è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Se è giusto punire le azioni o le parole che istigano alla violenza o ledono la dignità di una persona, non lo è però perseguire il dissenso o le critiche rispetto ai temi trattati nel disegno di legge che ormai porta il nome del deputato del L'esperienza comparatistica dimostra come norme analoghe a quelle contenute nel disegno di legge Zan abbiano portato all'incriminazione di persone per aver sostenuto che il matrimonio si fonda sull'unione di un uomo e di una donna o per essersi espressi criticamente verso alcuni atteggiamenti sul piano della sessualità, senza nessun legame con la violenza e con l'odio, e senza aver leso la dignità di alcuno. Anche il contenuto degli atti discriminatori e vietati non è definito in modo puntuale dal disegno di legge: così possono essere oggetto di sanzioni penali molte scelte delle persone che sono espressione di libertà protette dalla Costituzione, come quella di religione, di riunione, di associazione, di iniziativa economica ed altre. Molte sono le associazioni aperte solo a persone di uno o dell'altro sesso, che potrebbero veder minata la propria esistenza. Diverse possono essere le valutazioni sulle tematiche oggetto del provvedimento da parte delle confessioni religiose: pensiamo, ad esempio, alla nota della CEI a nome della Chiesa cattolica, ma anche alle scelte delle imprese di pubblicizzare i prodotti con immagini di coppie eterosessuali, e persino alle decisioni di alcuni artisti di non mettere il proprio estro e la propria creatività a servizio di determinate cause che potrebbero essere considerate ostili a qualche altra parte. Peraltro ci sono già esperienze di altri Paesi che hanno norme simili a quella che ora si vuole introdurre in Italia. Negli Stati Uniti un pasticcere è finito in tribunale per non aver voluto preparare una torta per celebrare una unione tra persone dello stesso sesso.

Per non parlare dei carcerati maschi che hanno chiesto di cambiare istituto penitenziario dichiarandosi di sesso opposto e la questione degli sportivi nati maschi che vogliono gareggiare con le sportive nate femmine. Pericolose appaiono anche le norme che utilizzano la scuola per promuovere ideologie di vario tipo, come quelle di genere, che vengono imposte per legge ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie e non invece il rispetto e l'amicizia tra i ragazzi che sono il fondamento della nostra istruzione. La disciplina ora sottoposta all'esame del Senato è anche fondata per molti aspetti su concetti assai ampi e indefiniti e rimette così la scelta dei comportamenti da punire alle valutazioni arbitrarie dei giudici, in contrasto con i principi di legalità, di tassatività e di certezza in materia penale garantiti dalla Costituzione repubblicana. L'articolo 4 del disegno di legge definisce addirittura, per renderli punibili, i comportamenti illegittimi, cioè garantiti dallo stesso ordinamento, qualora essi siano capaci a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori. Di fronte a tanti dubbi e a tante perplessità, anche molto autorevoli, perché sono stati espressi dal mondo accademico, da magistrati, da Presidenti di Consulta, il Senato anziché chiudersi avrebbe dovuto aprire un serio confronto tra le forze politiche e tra queste ultime e tutta la società civile sui temi oggetto del provvedimento. Siamo ancora alla discussione generale, ma l'augurio è che chi adesso si trova fermo ed immutabile sulle proprie posizioni si predisponga al dialogo, all'accoglimento di quelle modifiche che introducano una legge necessaria a tutelare determinati soggetti, ma che sia anche giusta e non discrimini tutti gli altri. *(Applausi)*. Mi hanno contattata nel 2016 in occasione dell'approvazione della legge sulle unioni civili, ringraziandomi per avergli restituito i loro diritti e la gioia di poter tornare a vivere nella propria terra, perché proprio grazie alla legge sulle coppie di fatto potevano finalmente scegliere di rientrare in Italia dopo essere stati per anni all'estero, per vivere qui liberamente il loro legame. Alcuni mesi fa, però, quei due ragazzi mi hanno scritto di nuovo raccontandomi che erano in procinto di ripartire perché in Italia non si sentono sicuri, sono stati più volte aggrediti per strada con insulti ed offese da parte di malintenzionati che li hanno assaliti dopo averli sorpresi mentre semplicemente si stavano baciando in pubblico. Purtroppo non sono i soli a subire simili soprusi: solo nell'ultimo anno, una persona LGBT su quattro ha subito minacce, violenze ed abusi omofobi sono aumentati in un anno del 9 numeri che da soli bastano a far capire quanto sia urgente approvare una legge che tuteli le persone dall'intolleranza, quell'intolleranza di chi non accetta che l'amore sia libero e personale. Solo trent'anni fa l'omosessualità rientrava ancora nell'elenco dell'Organizzazione mondiale della sanità tra le malattie mentali. Oggi l'omosessualità non è più considerata un disturbo, ma le persone LGBT in Italia, vale a dire lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e *transgender*, sono ancora esposti ad una condizione di vulnerabilità a causa di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale; discriminazioni che non solo sono scorrette dal punto di vista etico, ma che sono anche una violazione del principio di uguaglianza tutelato specificatamente dalla nostra Costituzione, che prevede che tutti i cittadini debbano essere messi nelle condizioni di esprimere la propria personalità e di vederla rispettata nel contesto sociale e collettivo. L'autonomia delle persone e la loro espressione nella società sono strettamente legate al rispetto e alla parità di trattamento che ricevono dagli altri ed è compito delle istituzioni, quindi è compito nostro, garantire l'individuo non solo come singolo ma anche nelle relazioni interpersonali e affettive ed è compito del legislatore lavorare per realizzare una società libera basata sul rispetto dei diritti e sulla valorizzazione delle persone, così da non permettere che l'identità o l'orientamento sessuale siano motivo di aggressioni di nessun tipo. Ecco perché è importante approvare questo disegno di legge, perché fa sì che ognuno sia libero di esprimere liberamente il proprio sé, senza subire limitazioni o violenze ingiuste ed intollerabili. Siamo, infatti, convinti dell'importanza della libertà personale anche nei sentimenti e nelle scelte di vita familiare. Il provvedimento ha inoltre il merito, grazie all'intervento della collega Lisa Noja alla Camera, di considerare atti discriminatori anche tutti quegli attacchi, quelle violenze e quegli atti di bullismo rivolti verso disabili, episodi che troppo spesso, ancora oggi, purtroppo rimangono impuniti. impuniti. Come Italia Viva, ci preme molto che questo provvedimento venga votato in tutti i passaggi salienti. Sia in Commissione che in Aula, abbiamo sempre sostenuto col nostro voto l'evolversi dell'*iter* del disegno di legge, ma temiamo che insistere ottusamente per la votazione in Aula, senza un accordo preliminare tra i Gruppi di maggioranza e senza un tentativo di mediazione tra le diverse forze politiche, significhi rischiare che il disegno di legge non vada in porto. Già ieri l'altro, con il voto sulle questioni pregiudiziali, abbiamo visto che il provvedimento è passato con appena 12 voti di scarto; e ieri ancora peggio, con appena un unico fragilissimo voto palese per scongiurare la questione Sono numeri, non supposizioni, che ci dicono che, ad ogni voto segreto, il rischio che il disegno di legge venga affossato sarà molto grande. Ecco perché continuiamo a confidare nel fatto che si possa ancora raggiungere un'intesa. Se fosse stata accolta la sintesi elaborata dal relatore, presidente Ostellari, che aveva sostanzialmente recepito *in toto* anche le nostre proposte emendative, adesso con certezza potremmo definitivamente approvare il provvedimento al Senato e potremmo blindarlo, con l'accordo politico di votarlo alla Camera nel giro di poche settimane ponendo la fiducia. grazie a modifiche che non sminuirebbero il senso del provvedimento, perché si tratta di formulazioni simili, estratte da un analogo disegno di legge, presentato sul medesimo argomento dal collega Scalfarotto. Proposte che erano già state condivise e sottoscritte dall'onorevole Zan ad inizio legislatura. Con questi nostri emendamenti, noi chiediamo di fare politica. Fare politica significa essere disposti a scendere a compromessi. Il muro contro muro non porta da nessuna parte. Bisogna sapere mediare per poter trovare punti di incontro che interpretino gli interessi dei cittadini e delle cittadine. Come Italia Viva alla Camera abbiamo approvato il testo attuale del disegno di legge Zan perché lì c'erano voti sufficienti. Oggi, però, se vogliamo portare a casa il risultato, dobbiamo confrontarci con i numeri del Senato e la realtà ci dice che i numeri al Senato, con alta probabilità, non saranno abbastanza. Ecco perché mi sento di rivolgere a mia volta un appello alle forze parlamentari riformiste e liberali: modifichiamo insieme il provvedimento. Sediamoci ancora attorno ad un tavolo e individuiamo quegli aspetti che ci consentano di perseguire un consenso ampio, tale da blindare la legge senza esporla a brutte sorprese. Il provvedimento è troppo importante per rischiare che decada nella anonimità di voti segreti. Sono tanti i colleghi che si riconoscono nell'idea di un'Italia moderna ed europea e di un Paese dove le libertà personali vengono riconosciute e tutelate. È a questi colleghi che mi rivolgo; a loro mando l'invito ad esprimersi a favore di alcune modifiche puntuali, che portino ad un più largo consenso e che ci consentano di trovare insieme un compromesso attraverso il quale approvare la legge senza intoppi. Questa legge è urgente, è necessaria. È una legge per una società orientata a domani ed esprime il bisogno di un ammodernamento sociale, per un salto in avanti che è opportuno che l'Italia compia. Noi di Italia Viva siamo convinti che non sia giusto fare delle battaglie fini a se stesse senza creare i presupposti per portare a casa il risultato. E riteniamo che non sia corretto nei confronti delle persone muoversi con l'unico obiettivo di guadagnare qualche *follower* in più, se poi i diritti si perdono per strada. Noi non siamo per una politica del lascia o raddoppia. A noi premono i risultati concreti. Siamo quelli delle unioni civili e siamo qui oggi per aggiungere un ulteriore tassello al percorso della parità dei diritti avviato con il nostro provvedimento nel 2016. Non ci piace doverci ritrovare in Aula a fare gli scongiuri, appesi all'incertezza di qualche voto di scarto. Da noi di Italia viva continua ad esserci un voto leale e costruttivo, in linea con quanto fatto fino ad ora. Ma siamo sicuri che l'atteggiamento del resto della maggioranza potrà dirsi altrettanto leale e trasparente? Se, come temiamo, nel corso di singoli voti segreti i numeri tradiranno questo provvedimento e lo faranno decadere, non ci si venga a dire che siamo stati noi di Italia Viva a farlo affossare. Noi voteremo convintamente a favore del disegno di legge, come abbiamo fatto in ogni passaggio fino a questo momento e invitiamo tutti a fare altrettanto, così che ci sia un consenso sufficiente per farlo passare, così che storie di aggressione come quelle a Pietro e a Valerio possano finalmente venire denunciate e condannate. Ma se vogliamo realmente cambiare questo Paese è ora di uscire dal vicolo cieco di posizioni teologiche e vedere come tutelare davvero gli interessi di tanti ragazzi e persone perbene che chiedono soltanto di potersi amare senza fare del male a nessuno. *(Applausi)*.

perché vedo che il dibattito gira intorno a totem ideologici, a surrogati di pensiero. Mi spiego

spero di sbagliare, ma temo di non sbagliare molto - dietro a questo provvedimento c'è un consueto atteggiamento di un certo pezzo di sinistra che, avendo nel tempo depauperato la portata del proprio pensiero ideologico sotto i colpi di un tatticismo esasperato (che, ad esempio, vede oggi il PD governare insieme alla Lega), è è costretta a surrogati di pensiero che deve blindare. Il pensiero della sinistra viene da un pensiero forte il quale non ho nulla da spartire, ma che rispetto profondamente, laddove ancora esiste, tant'è che rispetto quei colleghi che ancora nutrono quel pensiero e lo manifestano esplicitamente, concretamente e coerentemente. Gran parte della sinistra, però, questo pensiero se l'è giocato; la sbrindellato, l'ha perso dietro un percorso ipertattico per dover gestire il potere a tutti i costi, a tutti i costi, e gli ultimi dieci anni rispetto a questo sono assolutamente palesi, lampanti ed esaustivi. Di cosa c'è bisogno per aggregare? Di montare il nemico, di costruire il totem ideologico e, allora, a turno riscopriamo il pericolo del fascismo e l'intolleranza nei confronti del diverso.

Giustamente si pretende il rispetto per il diverso, ma secondo me è un'offesa anche definirlo tale perché per me, invece, non c'è niente di diverso in una persona che sceglie nella propria vita di fare ciò che vuole rimanendo nel lecito. Per me non c'è nulla di diverso quindi, non lo considero un diverso. Mi torna in mente il termine che conoscevamo da ragazzi «invertito». Lo ricordate? Per me è un offesa ovviamente ed è un'offesa anche dire che è un diverso. Per me non è un diverso; è un uguale, ma io sono per l'uguaglianza in partenza e, comunque, qui rischiamo di divagare. Quindi, di fronte a un testo che dovrebbe o vorrebbe tutelare il diverso, quale maggiore diversità va tutelata, se non quella del pensiero, quella di poter esprimere liberamente, tranquillamente e serenamente il proprio pensiero, anche quando è assolutamente incontrovertibile.

al di là delle donne, qualcuno possa procreare, questo passaggio, qualora sia inserito in una discussione dove c'è di mezzo un ragionamento che attiene all'orientamento sessuale - chiamiamolo così - può essere giudicato da un magistrato zelante come discriminante o istigatorio, perché lascia totale libertà di giudizio, senza mettere paletti o parametri. E vi garantisco che questo, alla prima sentenza, come è stato correttamente fatto notare da alcuni

o pretendereste che aprissimo con questo passaggio. Mi rifiuto però di pensare che ciò non possa essere compreso dai colleghi che ho di fronte e quindi

a prescindere da ogni altra considerazione logica, come quelle espresse dai colleghi di Forza Italia e della Lega e anche dai colleghi di Italia viva e di parte dei colleghi del PD, come nell'intervento di ieri dell'ex capogruppo, senatore Marcucci. Quindi, quando si va a tutti i costi, evidentemente non c'è nessuna possibilità di mediazione. Non la si vuole la mediazione, perché l'obiettivo politico non è tutelare il diverso, come voi lo chiamate, ma è costruirsi un abito ideologico e mentale, da poter propinare come surrogato ideologico a un elettorato ormai stanco, che non sa più cosa votare e perché votare. Perché un elettore oggi dovrebbe votare PD?

tattici sono esclusivamente necessari a ciò. In tutto questo, il problema è che ci vanno di mezzo diritti fondamentali assolutamente non negoziabili. Non è possibile comprimere la libertà di opinione e di giudizio, fino al punto di non poter dire cose assolutamente normali, come il fatto di poter dire che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Possiamo non essere d'accordo su questo: vivaddio se non siamo d'accordo su questo! Ci può essere una parte che dice che un bambino non ha bisogno di un padre e una madre, ma di due genitori che lo amano. Va bene, mi sta benissimo, ma voglio poterlo dire, voglio poterlo affermare liberamente ovunque che, secondo me, un bambino ha bisogno di un padre e di una madre e ne potrei dire altre 20 o 30 di queste cose. Ricordo a

per cui io una settimana decido di stare dentro il genere maschile e frequento gli spogliatoi dei maschi, poi,

*(FdI)*. Mi rifiuto di pensare che ci possa essere un'intelligenza che non percepisce l'assurdità di questo testo. Mi resta solo da considerare il tatticismo che c'è dietro;

resta per me motivo di preoccupazione quando vedo che in realtà semplicemente non ci si ascolta, perché si sta fuori. Quindi noi non ci facciamo carico delle argomentazioni degli altri, che la pensano diversamente da noi, e gli altri non hanno modo di assorbire nel dibattito parlamentare quelle argomentazioni che forse finora sono rimaste ai margini di una riflessione personale. Mi dispiace un po', ma questa è la prerogativa del dibattito in Assemblea, in cui ognuno parla, ma non c'è confronto immediato e diretto. Questo sembra consacrare posizioni diverse e non andare verso quella linea di mediazione, che avrebbe potuto essere l'obiettivo dominante di un lavoro in Commissione e che a mio avviso avrebbe potuto rappresentare davvero la possibilità di andare incontro a una capacità di raccogliere dubbi, paure, perplessità, ma anche desideri e aspettative di tutte le persone. Cosa registro io in questo momento? Registro positivamente una cosa: immagino tutte le famiglie che hanno figli omosessuali immagino tutti i ragazzi e tutte le ragazze omosessuali che da questo dibattito comunque traggono un elemento importante di speranza e di sicurezza. Non c'è nessuno che si opponga a loro, nessuno che contesti il loro orientamento e nessuno che vada rivendicando sanzioni nei confronti del loro comportamento. Io immagino che, dopo queste giornate, dopo tutto quanto la stampa ha detto e dopo tutto quello che appare nei telegiornali, un ragazzo possa andare con più semplicità a casa sua, dai propri genitori, e dire loro di essere omosessuale

Immagino che questa totale e assoluta trasversalità degli interventi, che riconoscono all'orientamento sessuale di ognuno, qualunque esso sia, il proprio diritto a esistere, si traduca di fatto, a livello personale in queste situazioni, nella maggiore di libertà di esprimersi, nella maggiore sicurezza di essere accolti e nella sostanziale speranza di poter costruire un percorso insieme.

Nello stesso tempo, immagino che a tante altre persone questa stessa impostazione e questa stessa riflessione dovrebbero far conquistare una maggiore pulcritudine nel linguaggio. Esiste la violenza fisica, che tutti noi conosciamo e sulla quale ognuno di noi si esprime negativamente; la violenza, qualunque essa sia, contro chiunque e per qualunque motivo, motivo, resta sempre la versione meno umana dell'uomo, quella biologicamente più vicina alla componente animale che ognuno di noi ha, quando, non avendo il bene della parola, soltanto la forza e la violenza determinano le scelte. Per noi non è così, però immagino che questo dibattito aiuti anche moltissimo le persone a curare il loro linguaggio, ad essere prudenti e consapevoli che le parole feriscono e che quindi non si possono utilizzare termini capaci di mortificare l'altro, a cui va riconosciuta la libertà di poter esistere nella complessità delle scelte affettive che ha inteso fare. Questa è già una conquista del presente dibattito: gli uni più prudenti nell'esprimere sempre e comunque il proprio pensiero, stando bene attenti che l'espressione del pensiero non rappresenti quella punta di violenza che umilia e mortifica l'altro; gli altri più convinti di una libertà di scelte che hanno fatto e della certezza che in questa inclusione saranno le proprie famiglie, a cominciare da queste, ad essere accoglienti.

di formulare ognuno le proprie scelte in una relazione che legittima gli uni e gli altri nelle proprie posizioni, che io stessa ho firmato il disegno di legge a prima firma della senatrice Licia Ronzulli. Si tratta, però, di un disegno di legge in cui il punto forte, rappresenta il cuore di tutto il dibattito, ribadisce questo rifiuto della violenza e quindi rilancia l'idea di una civiltà e di una civilizzazione che mi piace chiamare, come faceva Paolo VI, la civiltà dell'amore in senso profondo.

tutte le caratteristiche e la connotazione previste sotto il profilo anche della loro sessualità; proprio questo rispetto per la libertà suscita in molti di noi moltissime perplessità a che questa scelta libera abbia un coinvolgimento

anche quando parliamo del famoso articolo 7, che preoccupa nella misura in cui quella che dovrebbe essere un'indicazione all'inclusione, all'accoglienza e anche al rispetto reciproco possa tradursi in un indottrinamento.

in genere su questi argomenti dei diritti civili la società anglosassone è più avanti a noi. Quando dico più avanti a noi non intendo dire meglio di noi, ma semplicemente cronologicamente più avanti a noi: accade prima lì e poi qui.

Non è una paura sospesa per aria; è un'esperienza reale: sappiamo che accade prima lì e poi arriva qui, volenti o nolenti. La seconda cosa l'abbiamo vissuta tutti con i libri di testo che non sto qui a citare: è una forzatura dover dover considerare la diversità sessuale come un elemento intrinsecamente discriminante. Voglio citare i libri delle elementari con i pinguini, per non avere una madre e un padre, e mille esempi in cui si finisce con

comunque esiste un'azione forte, che è quella dell'educazione, che offre meccanismi di rinforzo. L'educazione precedente, di qualche decennio fa, aveva una serie di meccanismi di rinforzo all'identità di genere. Uso questa espressione intenzionalmente. Si cercava di coltivare nelle bambine la loro femminilità e nei maschi la loro mascolinità. Probabilmente si commettevano degli errori, ma vi era la consapevolezza che questa identità dovesse essere sostenuta attraverso meccanismi di educazione. È stata fatta una campagna quasi a tappeto per eliminare tutti i cosiddetti stereotipi di genere sul piano educativo, lasciando i bambini davanti, davvero, all'indeterminatezza del sé. Ciò non può essere assunto, in questo momento, come un'argomentazione a sostegno di questa teoria; piuttosto va preso atto, dal punto di vista educativo, che noi dobbiamo sostenere, nei modi, nei tempi, nelle circostanze, con i modelli, tutti quei processi che rafforzano nei ragazzi e nelle ragazze questa identità. Concludo, signor Presidente, e la ringrazio per questa manciata

Non voglio fare una profezia, ma voglio dirvi che non può passare, perché contiene al suo interno una serie di distorsioni reali. Lavoriamo su quei punti, perché abbiamo la possibilità di farlo; non lo faremo in Commissione, pazienza. Lo faremo con gli emendamenti,

Su questi emendamenti si gioca la vita della legge, se passa o no, e il messaggio forte che lanciamo ai ragazzi e alle ragazze della comunità LGBTQ+, ma anche a tutto il resto della società. Non abbiate paura: lo diciamo agli uni e agli altri. La nostra forza sarà la forza degli emendamenti e la nostra responsabilità sarà la responsabilità degli emendamenti.

sono profondamente contraria all'approvazione di questo disegno di legge, in particolare nei confronti di alcuni articoli. Penso che ai bambini non debba assolutamente essere trasmessa l'ideologia *gender*; spetta ai genitori educarli, non certo ad altri. Non siamo nell'ex Unione Sovietica, dove i bambini venivano tolti alle famiglie ed educati dal Partito. I vostri desideri non vanno confusi con i diritti: sono dei capricci ideologici che limitano le libertà degli altri e per questo mi opporrò con ogni mezzo lecito ad evitare una legge siffatta, che strangola la mia libertà e quella di chi mi ha eletto e che rappresento. I bimbi hanno diritto ad un padre e una madre. Quando sono grandi vogliono sapere perché la madre biologica li ha abbandonati e soffriranno moltissimo per tutta la vita. Non potete pretendere questo, con l'utero in affitto, pur di soddisfare i vostri desideri. Fate nascere i bimbi in maniera normale, senza dover pagare delle povere donne per farveli consegnare. Siamo arrivati alla deriva morale. Per non parlare della mancanza di qualsivoglia evidenza scientifica circa tutta la cinquantina di generi che sostenete esistere. Cosa volete insegnare ai bambini se non c'è alcuna base scientifica? È come se affermassi - scusate - che piovono patate e non acqua e minacciassi di portare in tribunale chiunque osi metterlo in dubbio. Penso che qualcuno abbia bisogno di tutele e supporto, ma questo senza creare danni ai bambini e limitare la libertà altrui. Non comprendo come una trentina di aggressioni annue, perlopiù verbali, nei confronti delle persone LGBT, possano costituire un'emergenza nazionale e motivo per approvare questo disegno di legge: ma per favore, dai, avete mai pensato alle donne italiane vittime quotidianamente di stupri da parte di stranieri, in particolare quelli di religione islamica e culture completamente diverse dalla nostra? Pensate a Pamela, fatta a pezzi e messa in due valigie, o a Desirée: questa è emergenza vera. O forse noi donne non abbiamo la stessa dignità degli LGBT? Per non parlare delle donne immigrate, sottoposte a mutilazioni o fatte sparire o costrette a sposarsi contro la loro volontà. Non ho sentito alcun difensore nei loro confronti o proporre qualche legge per tutelarle. Personalmente non ho alcuna fobia verso gli omosessuali e tutte le altre categorie LGBT; le considero proprio persone degne di rispetto. Sono esattamente come tutti, perciò vivano la loro vita come meglio gli garba, senza però limitare tutte le libertà degli altri. Soprattutto rispettino i bambini che hanno i loro diritti, senza operare forzature nel loro percorso formativo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento si soffermerà su alcuni aspetti paradossali che stanno caratterizzando questa discussione a un provvedimento riconosciuto importante da tutti, sul quale, viceversa, ancora l'altro giorno è stata posta una questione pregiudiziale di costituzionalità e ieri la questione sospensiva per tentare di bloccarlo. Il dibattito sul disegno di legge Zan sembra vertere su questioni di dettaglio, procedurali, di prassi parlamentare, sull'esagerata dilazione dei tempi o meno. Ce ne ha dato un saggio l'altro giorno il presidente Ostellari, rivendicando il ruolo del Senato, che non è chiamato a ratificare le deliberazioni della Camera dei deputati: giusto, corretto; non si capisce, però, l'atteggiamento ostruzionistico portato avanti in questi mesi dal Presidente della Commissione giustizia. Il senatore Renzi si è spinto ancora oltre: ha ricordato che lui era per l'abolizione del bicameralismo perfetto ma, dopo l'esito del *referendum*, è diventato un campione del ruolo specifico del Senato, il quale, in pochi giorni, può fare una mediazione che non è stata possibile in otto mesi. Non solo. Secondo Renzi, il Senato può dar vita a un patto tra le forze politiche per una rapida approvazione anche alla Camera dei deputati. In queste schermaglie tutte politiche sono assenti i contenuti del provvedimento oggetto del nostro dibattito; sono messe in sordina tesi e antitesi che invece hanno riempito in questi mesi le pagine dei giornali, ma che non hanno avuto modo di essere approfondite in quest'Assemblea. Tutti riconoscono che il disegno di legge Zan è importantissimo, che non deve avere un intestatario politico, che non può rischiare il voto segreto, ma che deve essere votato alla luce del sole, dal più ampio schieramento di forze in ossequio all'ampia maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Basta la volontà di entrare nel merito dei contenuti del disegno di legge Zan per capire, come è successo nel dibattito di questi due giorni, che il divario tra gli schieramenti politici è molto netto. Un grande filosofo della scolastica, Pietro Abelardo - mi viene in mente lui - constatato che su diverse questioni teologiche le sentenze dei padri della Chiesa erano spesso divergenti e qualche volta antitetiche, propose un metodo che sta ancora oggi alla base dell'insegnamento universitario: il metodo del *sic et non*, delle *quaestiones disputatae*, che portarono a quei quaderni *quodlibet*, fondamentali per la crescita e lo sviluppo del dibattito. Abelardo antepose al principio di autorità quello della ragione per venire a capo e prendere ragionevolmente partito su una tesi. Tutto il contrario, mi pare, di quanto si sta cercando di fare oggi in questo dibattito. Tra l'autorità del senatore Pillon, che contrappone la scienza all'antropologia, e quella del senatore Salvini, che proclama che all'interno di questo Senato non vi è alcun parlamentare che sostiene arcaiche discriminazioni di genere, non ci può essere mediazione. O rispetto alle affermazioni dell'autorità del presidente Ciriani, secondo il quale famiglia è unione tra uomo e donna in funzione della riproduzione c'è mediazione possibile rispetto all'autorità ancora del senatore Salvini, che accoglierebbe senza alcun problema a casa sua la compagna o il compagno di suo figlio? In politica la mediazione, lo sappiamo, è necessaria, ma essa non deve confondere le acque. Capisco che per un partito è meglio intestarsi una parte dei meriti per l'approvazione di un provvedimento riconosciuto come importantissimo, ma non sarebbe un disonore votare contro o astenersi quando vi sono ragionevoli dubbi. I *clerici vagantes*, per tornare al nostro Medioevo, alla fine della disamina delle varie e a volte opposte posizioni nel *sic et non* erano tenuti a prendere partito, che non era quello di una melassa impalpabile. Così si è affermato un metodo scientifico nelle nostre università. In caso contrario si inalbereranno vessilli identitari che alle *quaestiones* sostituiscono soltanto dei nomi. La ricaduta nominalistica non ci aiuta però a migliorare la conoscenza delle cose e, alla fine, se ci limitiamo ad essa, *nomina nuda tenemus*. Ad esempio, la parola genere dal latino *genus* e a partire dall'antico francese *genre*, diffusosi poi in inglese nella forma di *gender*, viene comunemente utilizzata per riferirsi a modelli di relazione, aspettative, vincoli e opportunità diverse tra uomini e donne. In questo si distingue dal sesso che invece rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile, quindi alla dimensione fisiologica. Orbene, intorno al sintagma identità di genere, si va sviluppando una divaricazione oltremodo pretestuosa. Parrebbe che a metterlo in legge significherebbe aprire le porte ad una definizione culturale della diversità, mentre non ammetterlo limiterebbe la definizione di legge a quella avente caratteri biologici. Non è assolutamente così. Il dato della giurisprudenza è ben altro. Già i dati normativi attuali, la Corte costituzionale con sentenza n. 221 del 2015 in materia di rettificazione giudiziale dell'attribuzione del sesso ha affermato che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n. 180 del 2017, nella quale ribadisce che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro un'espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. [**Presidenza del vice presidente LA Con la solita invasione di campo della giurisdizione nei confronti del Parlamento? Non sembra proprio. Le Corti dicono questo partendo proprio dalla parola «genere», che è già presente nelle varie leggi e decreti vigenti da vari anni nel nostro ordinamento, come la legge elettorale per la Camera e il decreto-legge n. 93 del 2013. Nulla di più facile, quindi, che la parola «genere» sia accettata nella mediazione cui il senatore Salvini accennava, senza che il collega Pillon battesse ciglio, una giurisprudenza coerente in pochi anni approdi ad applicare la legge Mancino anche all'identità di genere. Perché quindi tanto chiasso? Non è che sul rimandare o meno alla Camera il provvedimento si stanno per caso giocando partite, prove di tipo muscolare all'interno della maggioranza? Per concludere, sono assolutamente convinto che il disegno di legge Zan sia un provvedimento di civiltà, che ci aiuta a vivere in una società inclusiva, tollerante, rispettosa dei diritti di tutti, al di là e oltre i gruppi identitari che compongono la nostra variegata società.

della Santa Sede e alle lettere formali da parte della Chiesa apostolica in Italia e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in Italia stiamo andando avanti nell'illegalità, perché ci sono norme e documenti che sono diventati legge, come per l'appunto il Concordato, previsto dall'articolo 7 della Costituzione, e due delle Intese previste dall'articolo 8 della Costituzione, e vi sono dei passi formali previsti da quei Trattati, firmati dal Capo del Governo, che restano totalmente ignorati. Il Senato non è stato per nulla informato e tocca al Governo

questione dei diritti e delle discriminazioni delle persone omosessuali, transessuali e le altre che con sigle sempre più lunghe vengono menzionate a questo proposito,

che classificano gli atti omosessuali come reati e parecchi di questi prevedono anche la pena di morte per atti omosessuali. Ma di questi, a quanto pare, non interessa a nessuno dell'Assemblea che vuole il disegno di legge Zan a tutti i costi, presto, subito e senza cambiare una virgola. *(Applausi)*. A loro non interessa. Quando, poche settimane fa, è venuto il Ministro degli esteri iraniano in Italia, ho fatto dei comunicati e sono andato in piazza con la resistenza iraniana a dimostrare contro questo signore di un regime che esegue migliaia di sentenze di morte all'anno, che discrimina in modo gravissimo le donne, che finanzia il terrorismo e quant'altro, e che ha una legge piuttosto articolata sugli atti omosessuali. In essa intanto è prevista e praticata - non è prevista in teoria - la pena di morte,

non è islamica, c'è subito la pena di morte anche per la persona attiva. Diciamo che c'è una vasta articolazione. Ma anche di questo non interessa nulla; anzi, è stato ricevuto e non risulta dai resoconti ufficiali che il che il Ministro degli affari esteri abbia detto alcunché riguardo a queste "piccole" violazioni delle persone omosessuali che ci sono in Iran (piccole nel senso che le ammazzano e di conseguenza dopo non sono più discriminate). Però su questo non ho visto nessuno, ma neanche uno,

Voglio soffermarmi in particolare sull'articolo 8, che è stato un po' trascurato. L'articolo 8 dice che l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) - non mi risulta che l'omosessualità sia una razza, può essere tante cose ma non una razza - elabora una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e l'identità di genere, consultate le amministrazioni locali e - guarda caso - le associazioni LGBT (gli altri non interessano). Qualcuno chiederà chissà come sarà questa strategia; approviamo la legge e poi vediamo come sarà. Ma questa strategia già c'è ed è stata approvata addirittura alla fine del 2013 ed è pubblicata da allora sul sito dell'UNAR, che non è un'associazione privata, bensì un ufficio un ufficio del Dipartimento delle pari opportunità, che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Ed eccolo qui: quello che ho Su questo ho presentato un'interrogazione, fin da quando sono venuto a sapere di questo documento e del suo contenuto (nei primi mesi del 2014), ma non mi è mai stato risposto, e all'epoca facevo parte della maggioranza di Governo, così come ad oggi ne faccio parte. Anche in questa legislatura ho presentato al Ministro competente un'interrogazione per sapere se intendeva mantenere queste cose, ma non mi ha risposto e sono ampiamente passati i termini previsti dal Regolamento del Senato. Non penso proprio che in questi otto anni il contenuto possa essersi addolcito; semmai, viene accresciuto. Tanto è vero che il disegno di legge Scalfarotto della scorsa legislatura contro l'omofobia e quant'altro adesso è stato definito discriminatorio perché non include l'identità di genere; pertanto, semmai, questo documento sarà ulteriormente rafforzato. Cosa c'è in questo documento? C'è tantissimo: invito tutti coloro che sostengono il disegno di legge Zan, o comunque che si interessano di quello che succederà nel futuro, a leggerlo perché non è lunghissimo (sono una cinquantina di pagine),

cui si dicono tantissime cose e, in particolare, si dichiara che bisogna progettare percorsi innovativi di formazione in materia di educazione all'affettività che partano dai primi gradi dell'istruzione, - ripeto, dagli asili nido - e dalle scuole dell'infanzia a costruire un modello educativo inclusivo fondato sul rispetto delle differenze che costituisca una risorsa non solo per chi fa parte della comunità LGBT, ma per tutti i bambini. Dunque, dagli asili nido.

con tanto di riconoscimento di crediti formativi per chi vi partecipa, per cui è praticamente un obbligo o comunque un forte incentivo *(Applausi)*, con un particolare *focus* sul tema LGBT: lo sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente, l'educazione affettivo-sessuale, la conoscenza delle nuove realtà familiari. Quali sarebbero le nuove realtà familiari? Sarebbero le famiglie omogenitoriali, cioè coppie omosessuali con figli, dunque contro la legge, ma pazienza, tanto la legge poi si cambierà, alcuni giudici già ritengono di cambiarla. Un giudice ha detto persino che ogni tanto bisogna dare una spallata alla legge. Ma vorrei vedere cosa si direbbe di un generale che ogni tanto volesse dare una spallata alle istituzioni schierando i suoi carri armati. inoltre, che la formazione dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli studenti - figuriamoci - con il riconoscimento per entrambi di crediti formativi, ma anche a tutto il personale non docente e ai genitori. Si parla avvio di accordi di collaborazione con le associazioni LGBT e della valorizzazione dell'*expertise* - il testo è pieno di termini inglesi, perché a quanto pare l'italiano non è sufficientemente espressivo - delle associazioni LGBT in merito alla formazione e alla sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie.

Si va avanti dicendo tantissime altre cose e a pagina 42 di questo corposo testo c'è l'elenco delle associazioni con le quali si è collaborato e c'è una bella serie di associazioni LGBT, tra le quali il circolo culturale omosessuale Mario Mieli. Chi era Mario Mieli? lui è intitolato per l'appunto un circolo molto attivo, di cui ci sono anche dei filmati con delle *drag queen* che spiegano ai bambini il fatto che non devono limitare la propria sfera, pensare di essere maschi o di essere femmine, perché possono essere tutte e due, forse loro pensano di essere maschi ma in realtà sono femmine.

meno bello è quanto segue: «Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza». Un altro brano e concludo, perché è già fin troppo: «L'amore per Dio e il timore di Dio sono il risultato nevrotico di un amore per i genitori censurato dal tabù dell'incesto e da quello anti-omosessuale. Il desiderio erotico del bambino per il padre, il desiderio erotico della figlia per la madre, tutto si trasforma nevroticamente in adorazione di Dio, mentre l'esperienza magica dell'universo recondito... il conosci te stesso passano necessariamente attraverso l'omosessualità manifesta». Presentai a suo tempo un'interrogazione su questo,

la seguente: persone che intitolano il proprio circolo a un signore che ha scritto cose di questo genere che cosa insegnano ai bambini nelle scuole? Questa era la domanda: non c'è stata risposta.

condizionate con questa inclusività e dovranno esserci dei libri che portano in tale direzione. A proposito di libri,

visione. Sono due libri destinati ai bambini. Una recita: Milo si prepara per la nanna e poi ascolta la storia della sua nascita - ai bambini piace ascoltare le storie come le sue mamme si sono incontrate e amate e poi di come, per averlo, hanno chiesto aiuto un dottore che ha impiantato un semino nella pancia di una di loro. Il semino è diventato Milo, un bambino felice e amato. Siamo molto contenti che il bambino sia felice. mentre una volta si raccontava stupidamente della cicogna e dei cavoli, qui si racconta del dottore che mette un semino. Da dove viene quel semino? Viene da un uomo, che è il padre del bambino; bambino; bambino che avrebbe il diritto di averlo accanto a sé e di riceverne sostegno, tra l'altro anche economico. Invece no: è diventato un semino.

Da grandi, uno farà l'imprenditore - benissimo - e l'altro il pilota militare, molto bene. I due amici si sposeranno con una bella cerimonia festosa e con la benedizione delle loro mamme. Qui si insegna che l'amico del cuore o l'amica del cuore, per una bambina, è il tuo *partner* sessuale. Se non è così, vuol dire che è mancato qualcosa, che sei menomato. Ecco come andare a mettere in testa ai bambini idee di questo genere!

un video, girato durante un incontro organizzato dal professor Fedez, che è il nuovo intellettuale di riferimento per una certa sinistra. ci sono dei bambini e delle bambine che percepiscono il proprio genere fin da quando sono bambini; genere che è diverso dal loro sesso biologico. Ecco allora che bisogna aiutare quei bambini - e i genitori oggi sono molto più sensibili, fortunatamente, in questo - in un loro percorso di transizione, perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita. La presenza delle associazioni LGBT nelle scuole serve per andare dai bambini e dire loro: tu credevi di essere maschio, ma non è mica detto. Che ne sai? Ma che cosa ne sa un bambino se è maschio o femmina? O meglio: lo hanno sempre trattato da maschio, gli hanno anche spiegato le differenze tra un maschio le differenze tra un maschio e una femmina, perché evidentemente una femmina sa queste cose. Ma cosa gli si va a dire? Tu sei un bambino, ma forse sei una bambina? L'età dello sviluppo, l'età evolutiva, è già abbastanza complicata di

che vanno più nel dettaglio - ricordo che è scritto a livello molto alto perché è tra due Stati sovrani - mentre le intese con le chiese diverse da quella cattolica vanno più sul pratico, dicono non solo che i bambini che lo desiderano possono senza senza problemi essere esentati dalle ore di insegnamento della religione, ma che deve essere anche evitato l'insegnamento diffuso - così viene chiamato - di convinzioni religiose che non sono quelle del bambino o della sua famiglia. Qui come fai?

Quei gruppi o associazioni possono essere delle chiese, delle parrocchie, delle persone che si organizzano per fare una scuola a casa per evitare di essere indottrinati in questo modo. *(Applausi)*. Se sei tra gli organizzatori o i fondatori del gruppo, rischi fino a sei anni di reclusione. Come potete pensare che questa legge aggiunga diritti e non li tolga a nessuno? No: è una legge che contiene delle parti gravissime e che fa solo danno alle persone che, invece, dovrebbero essere protette che, invece, dovrebbero essere protette da un atteggiamento di tolleranza e accettazione generale. *(Applausi)*. Non bisogna insegnare solo ad accettare gli omosessuali e i transessuali;

perché non puoi rispettare gli altri se non rispetti prima te stesso. Tu rispetti te stesso se hai una dignità umana. La concezione del fatto che gli uomini sono uomini e donne e sono liberi di fare ciò che vogliono vogliono loro e non perché indotti da minorenni è fondamentale. Se tu non rispetti te stesso, non potrai rispettare gli altri. Se ti dicono che non sai quello che sei;

ti tolgono la dignità e, non avendo dignità, non rispetterai quella degli altri. Si va esattamente nella direzione opposta. *(Applausi)*. Bisogna insegnare ai bambini la loro cultura, la loro dignità, la loro personalità e rispettare quella degli altri. Questo è il rispetto. Questa legge, purtroppo, va in grandissima parte in direzione opposta.

il 4 novembre scorso, con una maggioranza diversa da quella che oggi è rappresentata in questo consesso. Premetto che la situazione non consente una grande libertà di scelta, nel senso che, se si propende per un prosieguo del dibattito, sia in Commissione che in proposte emendative, si rischia che il provvedimento venga definitivamente affossato e che quindi non vada avanti. L'alternativa appunto è quella di farlo passare così com'è.

questo sacrificio e la limitazione della libertà che ciascuno di noi si è dato siano alla fine utili e vadano nella direzione di tutelare veramente i soggetti LGBT, che hanno tutto il diritto di non essere discriminati e di vedere rappresentata la propria identità di genere all'interno di una di una società pienamente e ampiamente inclusiva, come quella che la Costituzione delinea e definisce chiaramente. Quello che però mi lascia estremamente perplessa è che

chiedo come mai tutti, sia di destra che di sinistra, si trovino d'accordo a sostenere e supportare una riforma della giustizia che cancellerà moltissimi reati, perché praticamente diventeranno impunibili a causa dell'improcedibilità dei vari gradi di giudizio, in appello e in Cassazione. che il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle e tutte le forze politiche che oggi stanno sostenendo il disegno di legge Zan - alle quali in questo momento mi ritengo vicina, perché penso sia giusto sostenere questo provvedimento, sebbene imperfetto

di fatto la possibilità della certezza della pena per tantissimi reati - figuriamoci per quelli in esame, che in questo provvedimento vengono delineati in maniera molto labile e difficile da dimostrare, perché l'onere della prova spetta sempre a chi accusa

punire in maniera rigorosa tutti i reati legati all'omofobia, sia sotto forma di aggravante

aspetto di vedere come procederà il dibattimento sulla riforma della giustizia. E mi attendo, proprio da quelle forze politiche che oggi stanno lavorando

a favore della certezza della pena e di una conclusione dei processi che renda giustizia non solo ai rei, ma anche alle vittime dei reati.

colleghi, ho letto il testo settario descritto dal senatore Malan e l'ho trovato inquietante in ogni singola riga. Comunque, Presidente e colleghi, questo provvedimento è servito più che altro per dare risalto a numerose personalità, più o meno note, che hanno preso posizione in merito e che si propongono come promotrici dell'acqua calda. La sessualità è una funzione intima, che va vissuta tra adulti consenzienti; non ha bisogno di Zan che suggerisca cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma l'alibi si regge sul fatto che le persone non etero subiscono maggiormente violenze rispetto alle persone etero. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Siamo sicuri che gran parte di quegli atti violenti siano esclusivamente messi in atto per ragioni di orientamento sessuale? Siamo così abituati ad ascoltare un tam tam assillante che ci impedisce la corretta valutazione dei casi. Proposte di legge selettive e fumose, come il disegno di legge n. 2005 e anche altre, non hanno senso di esistere, perché hanno finalità sottostanti implicite, che condannano e sanzionano la libertà di espressione. Il senso del nostro ruolo parlamentare non può essere banalizzato e incanalato in un'unica visione estrema, che vuole piegarsi al pietismo popolare, che è lo strumento che serve a gestire una situazione che si millanta tutela, ma che invece mira al controllo per omologare e a un consenso quasi automatico. Perché? Perché è più facile, signori. All'articolo 1, punto *d)*, si legge: «per identità di genere si intende l'identificazione percepita e e manifestata». Ma dal punto di vista giuridico cosa significa? Percepita come? Percepita quando, in quale contesto, in quale occasione? di legge, che presenta gravi criticità, favorisce l'ambiguità e ovviamente l'opportunismo di taluni. In pratica, se oggi dichiaro di percepirmi donna, posso partecipare a concorsi come quote rosa

A monte di un crimine come l'incitamento all'odio, ogni forma di odio, sia esso di tipo razziale, omofobo, misogino o culturale, ci sono dinamiche che il provvedimento nemmeno considera.

sono inquietanti. Si pretende di manipolare lo sviluppo dei bambini, ponendoli di fronte a tematiche che risultano essere poco pertinenti all'età e rischiano di minare le basi etiche della formazione primaria attribuendo alla scuola e agli insegnanti la responsabilità di affrontare un tema intuitivamente non condiviso da tutto il corpo docente, delegittimando di conseguenza la famiglia, famiglia, dove la figura educativa primaria è sempre stata e sempre rimarrà la figura genitoriale Anziché educare i bambini al rispetto per la vita, per tutte le vite, dalla più semplice alla più complessa, si vuole far loro credere che l'esperienza della realtà è una finzione, essendo l'umanità non biologica, ma oggetto di infinite, mutevoli mutevoli identità. Tutto questo è tradotto in un'età nella quale si va formando la percezione di sé in relazione al mondo che ci circonda.

Si svilisce l'istituto familiare e chi osa obiettare finisce sotto processo Tra i miei testi universitari c'era «Walden due» di Burrhus Skinner, uno psicologo comportamentalista, padre del condizionamento operante. Il condizionamento della società inizia plasmando la mente dei bambini. Della cosiddetta ideologia *gender,* alla alla quale il Papa ha riservato giudizi assai severi, si è capito che, anziché promuovere libertà di scelta e di azione, solleva profondi dubbi sulla facoltà di libera espressione. Chiunque potrà essere vittima di un procedimento penale, potrà essere sottoposto ad intercettazione o addirittura a misure cautelari. Un importante interrogativo rimane sull'autocertificazione della propria mutevole identità: se posso essere ciò che voglio e conta solo ciò che io io percepisco di me stesso, il resto diviene potenziale fonte di discriminazione nei miei confronti. Presidente, l'esito che ciascun magistrato darà, con la propria personale interpretazione, potrà essere solo un giudizio aleatorio, fatto di applicazioni disomogenee e arbitrarie. Come si potrà esercitare un dissenso rispetto a quella che diventa una legge di Stato? Lascia senza parola la pretesa di riscrivere, per legge, la natura umana e tutte le sue sfumature e sfaccettature, con una terminologia, per implementare un condizionamento che si esprime con parole come tutela tutela e libertà, ma che, in verità, impone una dottrina che non lascia alcun grado di libertà; una sentenza di condanna

sia importante e ritengo utile fare un punto della situazione, e non tanto da un punto di vista giuridico, legislativo e penale, perché i miei colleghi hanno spiegato e spiegheranno molto bene

molta animosità, furono molte le discussioni e credo sia importante ripartire proprio da quel momento. Vi sono infatti due aspetti che devono essere presi in considerazione. Il primo aspetto importante è capire chi era in quest'Aula e chi era fuori.

non c'è nessuno oggi, non c'era nessuno ieri e molto probabilmente non ci sarà nessuno neanche domani. *(Applausi)*. E questo - attenzione - avviene non perché il tema ovviamente non sia importante, ma probabilmente perché non è vero che i cittadini lo avvertono così di interesse, fermo restando che si tratta di un problema che dobbiamo e siamo in grado di risolvere. Probabilmente i cittadini non ritengono questo argomento prioritario.

che tutelano chi viene offeso con violenza, aspramente e duramente, a prescindere dal motivo per cui viene offeso, deriso, discriminato, allontanato e sbeffeggiato. In ognuno di detti casi, infatti, purtroppo discutibili, deprecabili e condannabili,

Non si comprende, quindi, il motivo per cui, andando a definire situazioni particolari, laddove evidentemente siamo tutti d'accordo in quest'Aula che una certa tipologia di reati debba necessariamente vedere un inasprimento delle pene, questo fatto non si traduca poi concretamente, in Commissione e in Assemblea, in una unanimità. Non si capisce perché non venga concesso avviso in maniera forzata - ma soprattutto alla Commissione, di formulare un testo che sia condiviso su un argomento sul quale alla fine siamo tutti d'accordo. Forse un motivo c'è. Il motivo - secondo me - è perché qualcuno qui dentro ritiene che i diritti civili stiano solo da una parte. Forse perché qualcuno ritiene, discriminando a sua volta, che solo una parte politica deve occuparsi di certi temi e soltanto a questa parte è delegata la tutela di certe persone. Ecco perché è importante partire da chi c'era fuori allora e da chi c'è fuori oggi, perché molto probabilmente stiamo sbagliando il nostro atteggiamento legislativo. Io personalmente ho una mia storia politica, breve breve o lunga, importante o meno che sia, che dura comunque da dieci anni, e come me l'hanno centinaia di migliaia di persone, alcune delle quali siedono in quest'Aula in questo momento. Insieme a tante persone abbiamo fatto un lungo percorso politico, che poi si è interrotto, ne è iniziato un altro, ma in tutto questo c'è un fatto fondamentale: nella mia carriera politica, ad esempio, nel MoVimento 5 Stelle, mai in dieci anni di attività politica - e sottolineo mai - è stato organizzato un gazebo o un banchetto a difesa dei diritti civili. Non è mai stata fatta una conferenza stampa a sostegno dei diritti civili. Perché dico questo? Forse perché i diritti civili non sono importanti? No, semplicemente perché, quando si fa politica, si alcuni argomenti. Io sono un esperto di tematiche aerospaziali e magari non mi interesso di giustizia; non ne capisco nulla e non mi interessa. La giustizia non è forse importante? Sì, ma non è il mio argomento. Questo era stato fatto. Era stata fatta una scelta ideologica, una scelta politica, e alcune tematiche - quelle che stiamo discutendo in questo momento - non facevano parte del DNA della mia ex forza politica. E ripeto non perché non fosse un tema importante, ma perché non ci interessava.

Sono molto preoccupato da chi dà sostegno oggi a un disegno di legge ovviamente liberticida, soprattutto da quelle persone che fino all'altro ieri erano completamente disinteressate al tema dei diritti civili. Detto questo, vorrei parlare di due aspetti tecnico-giuridici per quella che è la mia - seppur minima - competenza.

A me piacerebbe che nelle scuole entrassero soltanto gli insegnanti che hanno un contratto, che devono seguire un programma; vorrei che entrassero soltanto amministratori pubblici, autorità o le Forze dell'ordine in determinate cerimonie. Nessun altro, secondo me, dovrebbe essere titolato a entrare nelle scuole. Credo che lo Stato debba essere in grado di proteggere i propri figli da ingerenze esterne, da parte di persone non qualificate, ma scelte a caso nel mucchio semplicemente per convenienze politico-elettorali di facciata, di bandiera, che potrebbero essere veramente estremamente dannose. C'è, poi, un ultimo aspetto a quello che andremo, forse - speriamo di no - a raccontare ai ragazzi nelle scuole. Purtroppo, non c'è stata la possibilità di dibattere in Commissione, di fare tante audizioni su un tema così importante, su che cosa significa oggi l'attitudine sessuale, su che cos'è l'atteggiamento sessuale, quali sono le abitudini sessuali. Se avessimo avuto la possibilità di approfondire questo aspetto, forse avremmo capito che non tutto si può dire e raccontare, che non di tutto si può parlare con un bambino di sei, dieci,

Per questo motivo ho sposato la linea del nostro partito che è assolutamente di buon senso: è una linea logica, ma soprattutto è conforme alla nostra storia e alla cultura italiana. Non abbiamo bisogno di modelli europei. Non abbiamo bisogno di modelli transeuropei. Abbiamo bisogno di ricordarci quali sono le nostre tradizioni e qual è la nostra cultura. Questo possiamo farlo nel rispetto di tutti, lasciando liberi tutti i cittadini di amarsi e condividere la propria vita con chi si vuole, cercando però di rispettare ed equilibrare i diritti di tutti i cittadini.

Signor Presidente, Governo, colleghi, la discussione odierna verte su un argomento che probabilmente è uno dei più discussi in questo momento nei *social*, nei *media* e nell'ambito dei dibattiti pubblici. Sostanzialmente ne sta parlando chiunque, ne stanno parlando politici, artisti e *influencer*. Chiunque possa girare un video o scrivere un *post* in questo momento si è occupato o si occuperà a breve di questa discussione e non tanto perché effettivamente sia così sentita, ma perché si sta alimentando da quella che è diventata una contrapposizione ideologica. Il punto però per me non è questo, ma il seguente: di tutti questi soggetti che si stanno occupando del disegno quanti lo conoscono veramente? Quanti lo hanno letto? *(Applausi)*. Ecco perché nel mio intervento voglio riportare l'attenzione su quanto effettivamente è contenuto nell'articolato, quello che prevede esattamente il testo del disegno iniziando ovviamente dall'articolo 1, che contiene le definizioni. «Ai fini della presente legge: *a)* per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico». Per me dovrebbero coincidere, ma andiamo avanti. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso». Io ho una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti, ho una conoscenza empirica derivante da una competenza maturata in trenta anni di storia professionale e personale,

Alla lettera *c)* è previsto espressamente che «per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi». Questo è del tutto naturale, lo condivido e, quindi, andiamo avanti lettera *d)*: «per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione».

e transizione, nello stesso periodo. L'identità indica infatti, nel suo significato letterale, un rapporto di esatta eguaglianza; mentre invece la transizione indica un percorso, un *iter*, un passaggio da una situazione ad un'altra che sostanzialmente implica una dinamica di cambiamento, una evoluzione. Quindi o si parla di identità o si parla di transizione e non è una disquisizione meramente ideologica o di concetto, perché sostanzialmente poi, quando si andranno a valutare le applicazioni pratiche della legge, questa distinzione diventa fondamentale e - a mio avviso ma questa è una convinzione che ho da sempre e ritengo condivisa da tutto il mio Gruppo le norme devono essere chiare. Se infatti i concetti e le definizioni contenute nelle norme non sono chiare, poi si apre all'interpretazione e, inevitabilmente, l'interpretazione porta

L'oggettività sta nel fatto che i sessi sono due: non lo dice la Lega, non lo dico io e non lo dice solo la scienza, anche se, nel momento in cui due genitori vanno da un ginecologo a chiedere

perché mi mancherebbero quelle giuste per definire gli stessi concetti, dato che li condivido, ma semplicemente ritengo che sentir dire le stesse cose da chi, ideologicamente parlando, non è di certo della Lega, della coalizione di centrodestra, né vicino a me, può può consentire a qualcuno di capire che probabilmente si sta eccedendo in questa contrapposizione e strumentalizzazione di un *iter* di legge che, a mio avviso, avrebbe necessitato di maggior cautela. definito in maniera chiara e inequivocabile che ci sono sia sostenitori sia detrattori del provvedimento, cerchiamo di capire se potrebbero aver maggior ragione i primi o i secondi. Secondo i sostenitori della legge, qui non si parla di di violazione o di limitazione dei diritti di alcuni, ma dell'affermazione di quelli di altri; vediamo allora se è vero, continuando sempre però non in una disquisizione fisiologica, ma nella lettura della legge. Nello specifico, immediatamente dopo l'articolo 1, all'articolo 2 è previsto di aggiornare l'articolo 604-*bis* del codice penale: si tratta uno degli articoli che regolano i delitti contro l'eguaglianza e che prevedono che siano puniti. Quindi, non è vero che parliamo di introdurre diritti, perché, dopo le definizioni, prevediamo di introdurre punizioni; quindi, la tesi sostenuta da molti colleghi in Aula dello schieramento della sinistra, che

con una lunga elencazione delle fattispecie di pena, l'articolo 604-*bis* del codice penale, proponendo appunto di punire chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Quindi, quando dite di voler introdurre diritti, sostenete una cosa che è smentita dal testo del disegno di legge. Bisognerebbe poi approfondire la distinzione tra propaganda e istigazione, che è quella sottigliezza che consente a qualcuno di introdurre un alibi (perché, a mio avviso, di questo si tratta), con cui sostenere che non è vero che si va a limitare la libertà di espressione, tutelata dalla nostra Costituzione. Purtroppo il tempo per approfondire questo argomento non ce l'ho, quindi mi limito a fare una provocazione e una domanda. È vero che qui si va a punire solo l'istigazione e non la propaganda (che è del tutto legittima, perché, se lo sono le rappresentanze di coloro che si identificano in una parte e la vogliono espressa, evidentemente lo è anche la propaganda)? È vero? I colleghi in tanti esempi hanno dimostrato che non è vero, perché, dove vigono leggi simile a queste, i fatti dimostrano il contrario. Il tempo a mia disposizione sta scadendo, quindi mi soffermo in maniera brevissima su quello che, a mio avviso, è il motivo vero di questo disegno di legge. Nella totale mancanza di un'ideologia di sinistra - e lo dimostra anche l'intervento dell'onorevole Izzo di ieri - il centrosinistra sta cercando di ricompattare le fila e di definire gli schieramenti dicendo: o noi o voi, o contrari o favorevoli. È il motivo per cui la nostra apertura e la nostra mano tesa, l'intervento del nostro segretario Salvini - che voleva veramente tutelare i diritti di chi ha bisogno - e quelli del presidente Renzi e di tutti coloro che si sono dichiarati disponibili al confronto - su cui ha tentato un'importante sintesi anche il presidente presidente Ostellari - sono stati rifiutati. Quelle porte aperte sono state chiuse, perché l'interesse della sinistra non è tutelare queste persone, ma darsi un'identità precisa, di cui altrimenti sarebbe priva per la totale negazione di quelli che erano stati i valori fondanti di quella precisa parte politica. *(Applausi)*. In questo modo, signori, non si fanno gli interessi di queste persone.

Avrei sperato - ma vedo che non ci sono segni in questo senso - che dagli approfondimenti e dagli interventi di ciascuno potessero nascere comunque il dubbio e la volontà di approfondire e di capire la tesi dell'altro. Mi sembra invece che stia diventando un mero esercizio oratorio e basta. Diciamo che il progresso che speravo di vedere, ossia lavorare per migliorare il testo

approvato in un ramo del Parlamento non possa essere rivisto, migliorato o maggiormente condiviso. *(Applausi)*. La vostra rigidità è dettata esclusivamente dall'ideologia, perché dev'essere così e basta e la verità, evidentemente, ce l'avete solo voi. Oppure, come diceva il collega Pazzaglini, vi serve avere una bandiera da da piantare in cima alla montagna: è mio questo risultato e fa niente se ci saranno storture pericolose. Ve l'hanno detto i colleghi che sono intervenuti negli ultimi due giorni: le storture ci sono, eccome.

Qualunque sia il loro orientamento, sono persone. Dovremmo riflettere - e provo modestamente a farlo io - su un'emergenza ancora superiore. Alcuni colleghi hanno toccato il tema: il valore che dovrebbe essere alla base di tutto il nostro dibattito è il rispetto, perché in quello innanzitutto di se stessi e degli altri sta la nonviolenza sulle donne, sui bambini, sui disabili e sulle persone LGBT. Questa è l'emergenza che dobbiamo affrontare. Nelle scuole vediamo che è sempre più diffuso il bullismo, che sia cyberbullismo o che sia violenza fisica

A prescindere, c'è questo bisogno di violenza, ma soprattutto l'assenza, evidentemente, di un'educazione al rispetto. quindi, è che bisogna lavorare su questo. Forse non tutti sanno che nelle scuole e nei Comuni si cerca di affiancare le famiglie con un sostegno alla genitorialità, non per far lavorare qualche educatore o qualche psicologo, ma perché serve. Alla fine, il nucleo forte che

anche da adulti. Quando ci sono le grandi difficoltà, infatti, alla fine, le persone cercano nella famiglia la possibilità di resistere, di ripartire, di essere comprese e di affrontare nuovamente altre sfide.

che porterà l'ideologia a creare situazioni stranissime e davvero pericolose, perché, se è giustamente ribadito il pluralismo delle idee, poi però si aggiunge: «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Chi lo decide? È talmente labile e sottile quel confine, che si possono creare mostruosità.

È abbastanza inquietante pensare che un domani non potremo non dico insultare, perché quello non si deve fare, ma dire che la si pensa in modo diverso rispetto ad altri,

ad anni molto lontani, quando anch'io ero giovane e tutti eravamo appassionati di musica, di Lou Reed, di David Bowie e di tanti altri artisti.

Non confondiamo le idee. Volevo sottolineare un'altra cosa, che forse non tutti sanno. In questo modo, stiamo anche sminuendo un problema immenso, quello delle persone che realmente si trovano in un corpo che non sentono proprio e che arrivano

Tale percorso è tanto incredibilmente traumatico, doloroso e terribile, che alcune persone che arrivano alla transizione definitiva con il cambiamento fisico del sesso fisico del sesso - non succede raramente - sono talmente distrutte da questo passaggio, che hanno potuto legittimamente fare, che arrivano persino a togliersi la vita, perché l'identità e

colleghe e colleghi, parto con un principio. Sono convinto che la diversità in tutte le sue espressioni in natura costituisca sicuramente un valore sia per il genere umano, sia quando parliamo di differenti temperature o di campi gravitazionali. Insomma, la diversità è ciò che rende vivo il nostro universo. Passando all'argomento nello specifico e parlando anche di sviluppo psicosessuale, si tratta di un processo naturale, che riguarda ognuno di noi, e di un aspetto fondamentale della complessa natura umana, costituisce certamente la sfera più intima e quanto di più privato. È un processo psichico e fisico che ha origine con il concepimento, poi prosegue con lo sviluppo e con l'educazione. I greci parlavano di eros, Freud parlava di libido; si potrebbe parlare anche di istinto in generale semplificando, è chiaro a tutti che poi però devono intervenire delle regole sociali. In una comunità intervengono anche il senso del pudore e, naturalmente, le necessarie leggi. Oggi più che mai è necessario legiferare proprio per porre regole che sono state forse anche annientate dal modo di vivere in una società senza riferimenti, che un famoso sociologo definiva liquida

nella società in cui sono cresciuti tanti di noi, oggi presenti in quest'Aula, forse c'erano più riferimenti rispetto a quelli che ci sono oggi e credo che non sia un processo evolutivo. La sfera sessuale, con i relativi comportamenti, resta sempre, secondo me, l'ambito più intimo e strettamente privato di ognuno di noi, così come anche - tema assai diverso - l'orientamento religioso. Nessuno può permettersi di giudicare o discriminare il prossimo per l'orientamento sessuale, così come per quello religioso, perché fanno parte entrambi della nostra sfera intima e della nostra libertà. Il principio di base,

Soggetti a giudizio, semmai, devono essere le nostre attitudini lavorative e il nostro impegno nel lavoro. Pubblici sono le nostre relazioni sociali e i modi con i quali ci relazioniamo con il prossimo e con gli altri in generale.

tutto. È accaduto in questi giorni, in quest'Aula, che, a causa di una supponente superiorità di certe sinistre ideologie, si volesse evitare la legittima e dovuta discussione su argomenti assai delicati. Accade che venga proposto di votare una legge così com'è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento, come se il nostro ruolo e il nostro punto di vista fossero ritenuti non solo non utili, ma perfino nocivi. Un simile atteggiamento è certamente lesivo delle più elementari regole democratiche e costituzionali. Quello che abbiamo chiesto e stiamo chiedendo, soprattutto in un Governo di larga maggioranza, è proprio di rispettare le opinioni di tutti, ma così facendo, col dichiarato intento di tutelare i diritti dei cittadini di questo Paese, si è cercato di limitare la libertà di espressione di noi stessi legislatori. Mi pare che di leggi provenienti dalla Camera dei deputati discusse ed emendate ce ne siano state tante, così come tante sono quelle in discussione e in attesa di essere approvate, su temi che, per quella che è la mia opinione, ritengo assai importanti, soprattutto nel contesto in cui stiamo vivendo. Tornando alla nostra Costituzione a alla nostra cultura, mi pare che, quanto a quella virtù chiamata tolleranza, a quella virtù chiamata tolleranza, gli italiani non debbano prendere lezioni da nessuno. La discussione è assolutamente necessaria, proprio perché per tanti aspetti, dal punto di vista giuridico, il tema è complesso. L'agone nel quale siamo stati trascinati e i toni che ne derivano rischiano di non farci affrontare gli argomenti in maniera compiuta. Occorre discutere e dare risposte alle esigenze di ognuno, secondo i nostri saldi principi costituzionali. anziché del sesso degli angeli (come si suol dire), ci potremmo trovare a discutere delle loro identità di genere, e non e non sarebbe certo un processo evolutivo, soprattutto in un contesto nel quale abbiamo anche tanto altro da programmare (e sappiamo quanti argomenti urgenti ci sono in discussione in tutte le Commissioni).

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'istruzione, il Ministro del turismo e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

dell'istruzione* - Premesso che: da anni tra 9.000 e 13.000 docenti di ruolo, secondo quanto si apprende incrociando i dati ISTAT e del contratto collettivo nazionale integrativo, presentano domanda di trasferimento interprovinciale, che permetta loro di rientrare o avvicinarsi alla sede di provenienza; solo una minima percentuale di queste domande viene soddisfatta a causa di un meccanismo poco chiaro e poco efficiente di assegnazione; numerose sono le criticità in parte riferibili al contratto collettivo integrativo sono state depositate in Senato e presso il Parlamento europeo petizioni volte a richiedere riaperture del contratto integrativo e l'attuazione di "mobilità straordinaria", in quanto la situazione ad oggi appare penalizzante

il flusso di informazioni che dovrebbe avvenire tra SIDI (sistema informatizzato del Ministero) e l'INPS, secondo un ordine di priorità e tenendo conto dell'effettiva disponibilità dei posti destinati alla mobilità, avviene non rispettando una cronologia logica e consequenziale, tanto che l'INPS dovrebbe riuscire a comunicare al Ministero i dati riferiti ai pensionamenti del personale docente in anticipo rispetto alla scadenza della presentazione delle domande di mobilità e conseguentemente prima che il SIDI venga chiuso. Ciò non avviene, in quanto le pratiche dei pensionamenti vanno lavorate successivamente alla presentazione della domanda di mobilità; considerato che: il diritto alla mobilità dei docenti di ruolo ha carattere di priorità come sancito nel testo unico dell'istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all'art. 470, comma 1, così recita "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità (...) per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico"; risulterebbe si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versano i docenti fuori sede e quali iniziative urgenti intenda adottare per porvi rimedio, anche adoperandosi di concerto con il Ministro del lavoro

e che lo stesso contratto, all'articolo 8, disciplina la disponibilità dei posti ai fini della mobilità, ricordo che per l'anno scolastico 2021-2022, ferma restando la riserva del 50 per cento per le immissioni in ruolo, la parte restante dei posti è stata destinata per metà alla mobilità territoriale e per l'altra metà alla mobilità professionale. Ciò posto, concordo con lei rispetto all'esigenza avvertita anche dal Ministero di acquisire tempestivamente i dati sulle cessazioni dal servizio che costituiscono il presupposto per poter avviare correttamente le procedure di avvio dell'anno scolastico tra cui quelle di mobilità. A tal fine, l'Amministrazione opera in costante raccordo con l'INPS: il termine per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è condiviso con l'Istituto previdenziale e indicato nella circolare dei pensionamenti. Tale data è tenuta in considerazione per la predisposizione dell'ordinanza ministeriale sui trasferimenti che dispone la chiusura delle funzionalità del Sidi per l'elaborazione delle domande di mobilità solo dopo l'avvenuto passaggio dei flussi informatici sulla certificazione dei pensionamenti da parte dell'INPS. Tuttavia, come ben sa, le criticità da lei segnalate non discendono tanto da questo fattore, pur rilevante, quanto piuttosto dal tradizionale disallineamento, a livello territoriale, tra i posti vacanti e disponibili e le sedi di residenza dei nostri insegnanti. Per concorrere a soddisfare le istanze di molti docenti, il Governo ha voluto dare una prima significativa risposta con l'articolo 58 del decreto-legge sostegni-*bis* che, modificando l'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione e l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, ha ridotto da cinque a tre anni il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti nella sede di prima assegnazione. La nuova previsione tiene in equilibrio l'esigenza di garantire la continuità didattica nella comunità educante e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti ad avvicinarsi ai territori di origine. Difatti, senatrice Drago, si rende necessario garantire un equo contemperamento tra esigenze contrapposte: da un lato, le legittime aspirazioni dei docenti, come da lei rappresentante; dall'altro, la necessità di assicurare adeguata stabilità agli organici così da migliorare la qualità della didattica attraverso la continuità. Ciò proprio nell'interesse dei nostri studenti. Colgo l'occasione per sottolineare come per l'anno scolastico 2021-2022, a fronte di 87.454 domande di mobilità, quelle soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4 per cento del totale dei docenti che hanno partecipato alla procedura ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di quasi 7.000 spostamenti fuori Regione.

è legato anche al tempo riservato alle domande di mobilità: durante le vacanze pasquali, come ben sapete, in periodo Covid, i docenti avrebbero dovuto prenotare la consulenza da parte dei sindacati. Altre problematiche sono legate proprio al contratto collettivo nazionale integrativo: il terzo anno, che sarebbe il prossimo anno scolastico 2021-2022, abbiamo riservato solo il 25 per cento

che stabilisce che «le procedure informatizzate non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico». Stiamo contravvenendo e infossando il *moral welfare* di docenti che per la maggior parte sono donne; quindi, non stiamo assolutamente tenendo conto di diritti civili. Abbiamo famiglie assolutamente allo stremo delle forze da tutti i punti di vista, soprattutto da quello economico ma anche da quello dell'equilibrio psicofisico. che oggi non diventi semplicemente... Signor Presidente, egregio signor Ministro, a quaranta giorni circa dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 vorremmo sapere, noi parlamentari, ma lo vogliono sapere tutti i cittadini, a che punto siamo con il piano di ripartenza nelle scuole in sicurezza, soprattutto con attenzione a quello che è il discorso legato al reperimento di nuovi spazi e di nuove aule scolastiche. Vorremmo approfondire la questione legata ai docenti e sapere se davvero quest'anno scolastico avremo tutte le cattedre assegnate. Dall'altra parte, vorremmo sapere se sarà seguito il tema del tracciamento dei contagi con particolare attenzione magari anche alla gratuità dei tamponi o dei *test* salivari, che sono meno invasivi e che potrebbero andare molto bene

anche in relazione alla sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi, che è un elemento importante e di recente sono stati stanziati 200.000 euro proprio per il suo Ministero per andare in questa direzione nelle scuole. Immaginiamo però non siano sufficienti. Vogliamo sapere esattamente a che punto siamo, con estrema chiarezza perché sui giornali e sui *media* ne sentiamo un po' di tutti i colori, compresa

Quando negli scorsi mesi si è avuta la seconda ondata pandemica, abbiamo comunque tenuto i bambini e le bambine della primaria a scuola e abbiamo ridotto al minimo l'utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri. I dati recenti dell'Invalsi, quelli di ieri, dimostrano che questo nostro continuo insistere sulla presenza aveva ragione e noi lavoriamo e stiamo lavorando tutti per questo. Ricordo però che

per gli stessi fini, ulteriori 60 milioni sono stati destinati alle scuole paritarie. Per gli enti locali sono stati attribuiti altri 70 milioni per l'affitto di locali e noleggio di strutture temporanee per aumentare, come da lei augurato, il numero degli spazi dedicati alla didattica. lei sa, nel cosiddetto decreto sostegni-*bis* abbiamo richiesto ulteriori risorse per quanto riguarda gli incarichi temporanei per il personale ATA e per il personale docente.

sostegni-bisabbiamo stanziato 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e previsto la possibilità per gli uffici scolastici regionali di stipulare direttamente convenzioni con operatori economici esercenti il servizio di trasporto. Le scuole potranno accedere inoltre ad un fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti. Su questo rimangono attivi gli strumenti fondamentali che sono i tavoli prefettizi. Per quanto riguarda il piano vaccinale, credo che esso giochi un ruolo fondamentale. Come lei sa, siamo già molto avanti; per quanto riguarda il personale docente, siamo già ad un livello tale che ci permette di cominciare a considerare

degli interventi e quant'altro. Ci auguriamo che, visto che manca poco tempo all'inizio dell'anno scolastico, si vada in questa direzione. Sulla questione delle vaccinazioni - lo ribadiamo

ci muoveremmo con maggiore cautela. Forse è meglio potenziare, con gli strumenti che abbiamo messo in evidenza, il sistema scolastico per garantire sicurezza agli studenti ed evitare delle scelte che spingono in qualche maniera nella direzione dell'obbligo. Ai ragazzi no. Dobbiamo garantire loro la presenza a scuola in sicurezza, ma su questo tema - già glielo anticipiamo - la Lega, se il Governo dovesse andare in tale direzione, comunque farà la sua battaglia.

certamente saprà, i dati relativi al turismo non sono purtroppo incoraggianti: si parla di quasi 88 miliardi persi nel 2020 e purtroppo anche il 2021 non sembra dare importanti segnali di ripresa, neppure con le prenotazioni estive. Sappiamo infatti dalle stime fatte che molti italiani hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia proprio per supportare il nostro turismo, ma tutto questo non risulta ancora pienamente sufficiente. Il ruolo del turismo straniero sappiamo quanto sia prezioso nel nostro Paese e una delle ragioni, purtroppo, che ha comportato una diminuzione del turismo estero in Italia è dovuta al ritardo del *green pass* europeo che - come sappiamo - può essere concesso dopo la guarigione da Covid-19, dopo il completamento del ciclo vaccinale, dopo quindici giorni dalla prima dose o, infine, con un tampone negativo effettuato nelle quarantotto ore precedenti. E sappiamo essere anche uno strumento di vitale importanza per partecipare a eventi come banchetti, matrimoni, feste. Noi pensiamo quindi che, a fronte dell'importanza nevralgica che riveste il *green pass* nella vita di tutti noi, dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare che l'intera economia del Paese possa essere danneggiata ulteriormente dai malfunzionamenti o dai ritardi nell'aggiornamento della situazione vaccinale che molti cittadini hanno lamentato anche in questi giorni. Al contempo, abbiamo visto emergere nuove tendenze per le destinazioni di villeggiatura, le cosiddette destinazioni secondarie, e cioè quei borghi storici, spesso in lento abbandono, ma ricchi di storia e di tradizione. Proprio per questo, Ministro, le chiedo, al nome del Gruppo Italia Viva-PSI che rappresento, quali misure intenda adottare per facilitare la stagione estiva, anche per i borghi cosiddetti di seconda destinazione, e di farsi promotore nelle sedi governative di un'eventuale opposizione a nuove restrizioni, anche se sappiamo che purtroppo le varianti non stanno certamente aiutando. Dobbiamo scongiurare in tutti i modi che ci siano chiusure come quelle che abbiamo già vissuto in tempi precedenti.

l'ipotesi di ulteriori restrizioni nella stagione estiva, che ovviamente ci vede contrari. Quanto al primo tema, le cose più importanti che abbiamo fatto sono sostanzialmente due.

Lo dimostra il PIL: questo sarà il primo anno nella storia della Repubblica, a mia memoria, che troverà una Nota di aggiornamento al DEF con un PIL superiore alla previsione

complici tutta una serie di questioni tra cui il *green pass* europeo, ma anche e soprattutto la decisione di riaprire dei settori come quello della ristorazione: questo fa fatturare. L'unico sostegno vero è tornare a lavorare; il resto sono chiacchiere. Venendo alle altre questioni, abbiamo inserito tutta una serie di misure finanziarie: dei 5 miliardi circa che riguardano il settore, mi fermo a quelli specifici

serve la responsabilità di tutti e serve rispettare, per quanto possibile, tutte le regole che ci siamo posti, ma non è possibile pensare a ulteriori restrizioni. *(Applausi)*. Pensiamo a un settore Pensiamo a un settore come quello delle discoteche: anche qui applichiamo il buon senso. È meglio riaprire con le regole piuttosto che far finta di niente e avere

intervenire in replica la senatrice Sbrollini, va nella direzione che indicavo anche nell'introduzione del nostro *question time*. Infatti, per far ripartire la nostra economia bisogna partire dal turismo e lavorare tutti insieme nella stessa direzione affinché

sia uno strumento davvero importante. Penso che, da una parte, sarebbe opportuno valutare sicuramente quello che sta facendo la Francia in questo senso e, dall'altra

*(PD)*. Signora Ministro, è convinzione condivisa che il PNRR rappresenti un'occasione unica per avviare il rilancio del Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese. Abbiamo lavorato molto di concerto perché il PNRR mettesse a disposizione delle otto Regioni del Mezzogiorno risorse quantificate in almeno il 40 per cento delle risorse territorializzabili e, quindi, parliamo di circa 82 miliardi, incluso il Fondo nazionale complementare al PNRR. Questi sono dati contenuti in un'apposita tabella pubblicata dal Governo nel suo sito, in cui sono ripartiti e definiti tra le sei missioni gli 81,55 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. diversi organi di stampa ed emittenti televisive nei giorni scorsi hanno sollevato un allarme che ha avuto una grossa eco, soprattutto nel Mezzogiorno; un allarme sulla base di alcune rielaborazioni fatte da alcune università sul *dossier* elaborato dai servizi studi delle due Camere circa l'effettiva destinazione al Mezzogiorno delle risorse del PNRR: si lamenta che quasi 35 miliardi su 82 abbiano effettiva destinazione territoriale al Sud, mentre per gli altri la destinazione territoriale sarebbe rimessa a scelte successive ancora non note. Considerato che la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione dell'intero PNRR e la mancanza di chiarezza sul punto della localizzazione territoriale degli interventi rischia di alimentare preoccupazioni e incertezze nei cittadini del Mezzogiorno, sono qui a chiederle se corrisponda al vero che gli 81,55 miliardi destinati al Mezzogiorno siano realmente tanti e non solo 35 e quale sia, in concreto, la quota esatta di risorse ripartita nelle singole missioni e nelle singole componenti; sia la quota a valere sulle risorse a fondo perduto e quale sui prestiti. Con queste domande, signora Ministra, conoscendo peraltro la sua sensibilità, le chiedo di rassicurarci e rassicurare il Mezzogiorno. Non è una questione di campanile:

la riduzione dei divari territoriali è uno degli obiettivi fondanti - come lei ha ricordato - del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie agli investimenti che abbiamo programmato e indirizzato al Mezzogiorno, per la prima volta dal Dopoguerra ad oggi, si produrrà una significativa convergenza delle due aree del Paese con una crescita del prodotto interno lordo del Sud superiore rispetto a quella del resto del Paese. L'impatto di investimenti e risorse produrrà una crescita al Sud del 24 per cento a fronte di una media nazionale del 15 per cento e una crescita dell'occupazione femminile giovanile rispettivamente del 5,5 per cento e del 4,9 per cento. L'obiettivo di investire almeno 82 miliardi di euro del PNRR nei territori del Mezzogiorno non è una promessa o un impegno generico, ma è il frutto di un attento lavoro di analisi, missione per missione, componente per componente, linea di intervento per linea di intervento, che abbiamo realizzato con gli uffici del MEF e delle altre amministrazioni competenti. L'importo finale dell'analisi, il famoso 40 per cento, è un risultato credibile e robusto. Non lo abbiamo detto noi, ma lo hanno detto gli stessi uffici della Commissione europea che, in fase di approvazione del PNRR, sulla base delle verifiche, delle simulazioni e dei controlli condotti, hanno confermato l'avvenuta assegnazione al Sud di una quota di risorse non inferiore al 40 per cento degli investimenti. È chiaro che raggiungeremo quest'obiettivo a due condizioni: che investimenti e riforme siano effettivamente realizzati nelle forme e nei modi che abbiamo puntualmente stimato e che saremo in grado, come sistema Paese, di accompagnare gli enti territoriali meridionali a progettare e a partecipare ai molti i bandi di gara previsti dal PNRR. Per sostenere questo enorme sforzo non ci siamo limitati soltanto alla fase di programmazione, che di per se è stato complicato realizzare in sole otto settimane, ma stiamo già lavorando concretamente alle attività di attuazione e monitoraggio della quota Sud. Stiamo per presentare un emendamento al decreto-legge *governance* per garantire che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR assicurino in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi, l'allocazione alle Regioni meridionali di almeno il 40 per cento delle risorse. Questo implica che, oltre agli interventi infrastrutturali già esplicitamente destinati al Mezzogiorno, almeno il 40 per cento delle risorse allocabile tramite bandi sia indirizzato al Sud. È un vero e proprio vincolo di destinazione territoriale fissato con una norma; le risorse ci sono e oggi ci sono anche gli strumenti di tutela della loro effettiva destinazione territoriale. In conclusione, Presidente, spero che le tante discussioni e polemiche dei mesi e delle settimane scorse, le giuste preoccupazioni ma anche le strumentalizzazioni - incomprensibili per il momento straordinario che stiamo vivendo, che impone a tutti di lavorare per costruire e migliorare anziché alimentare sfiducia - lascino ora il passo a un impegno comune e condiviso. *(PD)*. Signora Ministro, la ringrazio delle rassicurazioni e anche degli impegni che ha voluto qui ribadirci per sostenere

quello di offrire, anche nel Mezzogiorno, servizi, infrastrutture e diritti universali alla stessa stregua delle altre aree del Paese. Dobbiamo accompagnare questo sforzo e, per farlo,

se non si interverrà in questi termini rischieremo, con semplici bandi, che le amministrazioni più attrezzate continuino a drenare più risorse delle altre. Per questo mi dichiaro

*(FIBP-UDC)*. Gentile Ministro, le risorse per il Sud previste dal pacchetto Next generation EU, unitamente a tutte quelle risorse già previste dai fondi strutturali e dai fondi di sviluppo e coesione, sono ingentissime e hanno lo scopo, oggi, di colmare quel differenziale economico che c'è tra le aree del Mezzogiorno d'Italia e anche il resto del Paese, del Paese, compresa l'intera Europa. Il PNRR - lo abbiamo detto poc'anzi - attribuisce al Mezzogiorno d'Italia 82 miliardi di euro, che sono il 40 per cento di tutte le risorse territorializzate, e cioè che hanno una specifica destinazione sui nostri territori. Si apre, quindi, per il Paese una fase una nuova fase di convergenza tra le aree del Mezzogiorno d'Italia, quelle del Centro-Nord d'Italia, all'unico scopo indispensabile e importante dello sviluppo dell'intero Paese. Gli ultimi dieci anni, con un periodo di riferimento che va dal 2008 al 2018, non sono stati importanti per il Mezzogiorno d'Italia; al contrario, abbiamo assistito ad una spesa pubblica soprattutto per investimenti che si è ridotta notevolmente, anzi si è dimezzata e, prendendo questo periodo di riferimento, passiamo da una spesa pubblica di circa

infrastrutture fisiche, in infrastrutture digitali, in energia sostenibile, in edilizia residenziale pubblica, in rigenerazione delle aree urbane, ma soprattutto nei servizi alla persona. È quindi un'occasione importante. Individuata questa massa di risorse così importante, abbiamo la necessità di garantire

Ministro, qual è l'intenzione politica del Ministero per utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse e soprattutto se nell'ambito della normativa stessa si possono prevedere delle iniziative per evitare l'inerzia soprattutto delle pubbliche amministrazioni e, quindi, spendere bene tutte le risorse che abbiamo a disposizione in un momento storico così importante per il nostro Paese.

delle problematiche connesse all'effettiva capacità delle amministrazioni pubbliche responsabili di realizzare i piani, i programmi e gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, ovvero di utilizzare efficacemente il Fondo nazionale per le politiche di coesione. Come ricordato dall'onorevole interrogante, i prossimi anni costituiranno un difficile banco di prova perché ai fondi strutturali e nazionali si aggiungeranno le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo contesto, allo scopo di innalzare e rafforzare la capacità di assorbimento e garantire il rispetto dei tempi ai quali i finanziamenti sono agganciati, ho ritenuto opportuno rafforzare il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale. A tal fine, nell'ambito del decreto-legge cosiddetto *governance* e semplificazioni abbiamo lavorato per introdurre significative modifiche normative che affidano all'Agenzia per la coesione territoriale nuovi poteri in tema di *governance*, oltre quelli già previsti con riguardo all'attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e sostegno della politica di coesione. In primo luogo, è stato attribuito all'Agenzia l'esercizio del potere sostitutivo rispetto alle amministrazioni pubbliche il cui ritardo o inadempimento nell'attuazione dei programmi finanziati con i fondi strutturali può determinare il concreto rischio di definanziamento. Al fine di scongiurare questa ipotesi è ora previsto che, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione dei suddetti interventi, i poteri sostitutivi possano essere esercitati, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per il Sud e per la coesione territoriale, in quanto Ministro delegato per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, inoltre, può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi, considerata, peraltro, la specifica competenza tecnica di cui la stessa è dotata. Infine, sono state ulteriormente rafforzate le modalità di esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica degli obiettivi dei programmi finanziati dall'Unione europea o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. È adesso possibile che questi poteri possono essere esercitati, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale. Credo che questo sistema possa essere efficace per scongiurare il rischio di ritardi o, peggio, di definanziamento degli interventi.

Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, il PNRR stabilisce che al Sud andrà il 40 per cento dei fondi territorializzabili, ossia circa 82 miliardi. L'abbiamo detto poc'anzi. Tuttavia, in data 6 luglio «Il Mattino» ha pubblicato un articolo a firma del professor Gianfranco Viesti

Il professor Viesti ritiene che, sommando gli stanziamenti di ciascuna delle linee di intervento destinate al Meridione, risultano impegnati soltanto 22 miliardi di euro, anche se è altamente probabile che almeno altri 13 miliardi di euro saranno poi spesi nel Mezzogiorno in particolare, in alcune linee di intervento si trova una precisa indicazione della localizzazione territoriale della spesa, mentre in molte altre no. Questo non significa affatto che al Sud andranno solo 35 miliardi di euro, ma che solo questi sono garantiti con certezza. Infine, relativamente alle risorse non territorializzabili, nell'articolo di stampa ci si chiede dove andranno a finire le risorse, assolutamente maggioritarie, per le quali non vi è una allocazione territoriale predefinita, sostenendo che molto probabilmente finiranno in parte dove l'economia è più forte e ci sarà maggior "tiraggio" delle misure. In parte, conclude l'articolo, l'esito dipenderà dai contenuti delle norme attuative di riparto che verranno stabilite dai vari Ministeri che hanno la responsabilità e, in parte rilevante, dipenderà però dall'esito dei bandi che essi predisporranno, proprio per allocare su base competitiva le risorse tra i diversi beneficiari e, ancora, dai criteri che sempre i Ministeri definiranno per questi bandi. Quindi, signor Ministro, le chiedo se quanto riportato dalla stampa corrisponde al vero, se effettivamente risultano presenti nelle singole misure di spesa appena 35,3 miliardi di euro per il Sud, che ripeto sono pari al 16 per cento degli stanziamenti totali, quali siano i motivi per cui solo in alcune linee di intervento del Piano sia presente una precisa indicazione della localizzazione territoriale della spesa, quali siano le modalità attraverso cui verranno stabiliti i riparti delle risorse prive di una allocazione territoriale predefinita e, infine, se riguardo alle risorse non territorializzabili, intenda istituire sistemi di monitoraggio e informazione ai cittadini (*open data*) sui contenuti delle norme attuative di riparto e sui criteri di riparto previsti dai bandi, al fine di garantire il rispetto dell'equità territoriale.

a differenza dei fondi strutturali, non prevedevano e non prevedono alcun vincolo di destinazione regionale. Quindi, quando si dice che la Commissione europea ha imposto agli Stati dei parametri quantitativi da rispettare, si dice un'inesattezza. La Commissione chiede agli Stati membri di colmare i divari territoriali e la scelta del Governo, fin dalla fase di definizione del PNRR, è stata proprio quella di garantire che una parte rilevante e definita delle risorse fosse destinata al Sud, nella consapevolezza che l'obiettivo prioritario da realizzare fosse proprio quello di ridurre i divari territoriali, ma anche, naturalmente, di genere e generazionali. Quindi l'obiettivo solo trasversale del Piano, come era definito nella precedente versione del lavoro la riduzione del divario territoriale, è diventato un obiettivo centrale. La quota Sud del Piano e del fondo complementare è stata resa esplicita

lavoro così credibile e attendibile, che è stato ritenuto tale dalla Commissione europea, che lo ha incluso nella relazione di accompagnamento al parere favorevole espresso nei confronti del nostro piano. È evidente che le linee di intervento sono tra loro estremamente eterogenee. Ci sono interventi infrastrutturali definiti e geograficamente collocati, per i quali il riparto è immediato, soprattutto ad una prima lettura semplificata. Ci sono misure ad assorbimento come il superbonus, per i quali addirittura abbiamo usato criteri di riparto molto prudenziali, sulla base dei dati storici. Per esempio, per il superbonus si è stimato appena il 9 per cento al Sud, non tenendo nemmeno conto degli interventi di semplificazione, che potranno migliorare l'attrattività, introdotti nel decreto-legge semplificazioni. Ci sono infine misure a bando, per le quali si sono usati calcoli di riparto basati sulle esigenze, sui fabbisogni, sui divari e sulla capacità progettuale. Sui bandi si concentra l'attenzione del Governo. Come ho già detto prima, stiamo per inserire nel decreto-legge *governance* una disposizione per fissare normativamente il vincolo di riparto territoriale degli investimenti, a garanzia della percentuale del 40 per cento. L'assegnazione delle risorse sarà accompagnata da un monitoraggio puntuale dell'effettiva localizzazione degli interventi, svolto al massimo livello dalla cabina di regia, deputata insieme alla struttura centrale tecnica e a quella di missione presso il MEF, alle funzioni di verifica e controllo della destinazione territoriale. In caso di scostamento è prevista l'adozione di misure compensative e correttive. Quindi le risorse ci sono e ci sono anche gli strumenti per garantirne la corretta allocazione territoriale. Tuttavia io non mi ritengo completamente soddisfatta, anche alla luce di alcune sue dichiarazioni che ha fatto a mezzo stampa, in cui ha definito lo studio del professor Viesti un approccio tra l'ideologico e il ragionieristico. Tutelare l'equità territoriale vuol dire rispettare la Costituzione e non ideologizzare. ideologizzare. Il Parlamento esige proprio una quantificazione ben precisa dell'allocazione territoriale degli importi del PNRR. La mia interrogazione verte su una sola parola: certezza. certezza. Analizzando le 187 misure previste dal PNRR e dal fondo complementare, soltanto 61 prevedono certezza e precisano la quantificazione degli investimenti nel Sud. Laddove poi - come ha detto lei - non c'è indirizzo di allocazione territoriale, il reparto verrà effettuato soprattutto tramite la pubblicazione dei bandi; per questo motivo bisognerà prestare la massima attenzione a tutti quegli indicatori e a tutti quei criteri che troppo spesso hanno favorito soltanto alcuni contesti territoriali. Per questo motivo io avrei auspicato che il documento recante peso, percentuale e ammontare degli investimenti nel Mezzogiorno per ciascuna delle sei missioni fosse pubblicato anche nella versione ufficiale del PNRR e non soltanto sul sito del suo Ministero. Infine, apprendo con piacere che sta lavorando a un sistema di monitoraggio del rispetto della destinazione territoriale e non posso che plaudere a tale iniziativa, che dà seguito a quanto previsto da un mio emendamento al decreto fondo complementare, che obbliga il suo Ministero a presentare annualmente alle Camere, fino alla completa realizzazione del PNRR, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal decreto, anche sulla base del sistema di monitoraggio. Il Parlamento, signora Ministra, non chiede atti di fede incondizionata, ma certezze. Ovviamente abbiamo ancora fiducia nel Governo, ma auspichiamo che possa smentire con i fatti le preoccupazioni avanzate da uno studio ideologico e ragionieristico nell'interesse del popolo italiano.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Parlamento europeo ha riconosciuto la salute sessuale e riproduttiva tra i diritti umani. Nel testo approvato pochi giorni fa si afferma che i diritti alla salute, in particolare i diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sono diritti fondamentali delle donne, che dovrebbero essere rafforzati e che non possono essere in alcun modo indeboliti o revocati. Una decisione, quella presa, che va nella direzione di almeno tre degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: garantire una vita sana e promuovere il benessere e garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva per raggiungere l'uguaglianza di genere rientrano anche nelle azioni volte a creare una società pacifica e più inclusiva a tutti i livelli. Le violazioni della salute sessuale e riproduttiva delle donne costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e ostacolano il progresso verso la parità di genere. Ecco perché ora i Paesi dell'Unione europea dovranno garantire l'accesso a un'ampia gamma di servizi di alta qualità, completi e accessibili, nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti rimuovere tutte le barriere giuridiche, politiche, finanziarie e di altro tipo che impediscono il pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per tutte le persone. Nel testo si esortano gli Stati membri ad assicurare l'accesso universale all'aborto sicuro e legale e a garantire che l'aborto su richiesta sia legale nelle prime fasi nelle prime fasi della gravidanza, soprattutto se la salute della persona incinta è in pericolo. Non è una novità che alcuni Stati membri dell'Unione europea applicano leggi fortemente restrittive, che vietano o rendono difficilmente accessibile l'aborto, costringendo le donne a ricorrere all'aborto clandestino, a recarsi in altri Paesi o a portare a termine la gravidanza contro la loro libertà. Ciò costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere. Anche per l'Italia è arrivato il momento di adeguarsi alle direttive europee in fatto di

ministro Speranza e ai Presidenti di Regione, in particolare modo del Piemonte, dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e della Calabria, per dire che è giunto il momento di ripristinare i servizi alle donne, sia nei consultori sia negli ospedali. Le donne non sono persone di serie B, ma hanno diritto di avere accesso ai servizi che tutelino la loro salute sessuale e riproduttiva in piena libertà, come prevede la legge n. 194 del 1978 *(Applausi)*.

della morte di un giovane napoletano, Mario Paciolla, e un silenzio assordante avvolge dopo un anno la morte di questo ragazzo che partecipava ad una missione di pace per conto dell'ONU in Colombia. Mario Paciolla aveva trentatré anni quando, un anno fa, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di San Vicente del Caguan. Sappiamo che è stato trovato nella sua casa, appeso a un lenzuolo bianco e con tagli ai polsi. Non conosciamo ancora la verità, non sappiamo nulla di questo caso: è stato un suicidio o si è trattato di un omicidio? Se stato un omicidio, perché Mario Paciolla è stato ucciso? Colleghe e colleghi, Presidente, ricorderete tutti che all'epoca abbiamo interrogato in quest'Aula il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e che egli si è impegnato a fare pressione sull'ONU, sulle autorità colombiane, chiedendo la loro collaborazione per le indagini. Ma la sensazione un anno dopo è di una cortina oltre la quale non si riesce ad andare. Questa lunga attesa di dodici mesi ci sembra un'eternità. Non si sa nulla neppure sull'esito dell'autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Roma. È giunto il momento che la magistratura italiana renda pubblici i risultati dell'esame autoptico. I familiari e gli amici di Mario hanno il diritto di conoscere la verità, ma anche il nostro Paese deve sapere cosa è successo quel 15 luglio di un anno fa. Il caso Paciolla non può e non deve essere considerato un caso di serie B. Sappiamo che Mario era impaurito: ce lo racconta la madre che lo sentì al telefono poco prima di morire. Sappiamo anche che la scena del crimine fu alterata, pulita, e sullo sfondo c'è qualcosa che non convince e che riguarda proprio la missione ONU della quale faceva parte. Per questo mi è sembrato doveroso ricordare Mario Paciolla. Abbiamo bisogno tutti che si faccia chiarezza. Tutti noi ci sentiamo prigionieri di questo silenzio, impotenti di fronte al silenzio

semiaperta, ha strappato alla signora fede e orecchini, l'ha svestita e stuprata. Ovviamente la signora, nonostante una simile violazione, è riuscita a dare indicazioni e a fare arrestare il suo

nigeriano senza fissa dimora, con precedenti e con una domanda di protezione respinta. Si chiama Destiny Dike, persona che non doveva essere in Italia. Si tratta di due episodi inquietanti. Io penso che nessuno dovrebbe subire uno stupro. Fa orrore pensare a quanto accaduto a donne anziane, per quanto in gamba. Anche la seconda signora è riuscita a dare indicazioni così precise che il ventiseienne è stato arrestato poco dopo. dopo. L'urgenza è trovare il modo per fare prevenzione. C'è un'unica prevenzione, che è non avere

ma la cosa più facile che può avvenire è che vengano inserite nella criminalità organizzata, oppure vivano di espedienti e quindi delinquano abitualmente. Chi viene Chi viene nel nostro Paese deve seguire le regole. Invito il ministro Lamorgese a pensare a una politica che protegga i nostri cittadini,

lo si sa *a priori*, perché hanno la fedina penale sporca - non deve né venire né rimanere in Italia. Questo vuol dire fare prevenzione, non vuol dire essere cattivi. Noi dobbiamo difendere soprattutto le persone fragili, che sono anche le due signore che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

Grazie,